anche nei prossimi giorni, un risvolto di natura nazionale e forse anche - diciamo noi - di natura internazionale. Mi riferisco alla vicenda della richiesta di condanna a sei anni nei confronti di Matteo Salvini con

Anzi, noi abbiamo pieno rispetto sia dell'indipendenza della magistratura che anche del suo operato. Partiamo da questo presupposto. Consideriamo, però, ed è questo quello che vogliamo portare oggi all'attenzione dell'Aula,

la prassi in questi casi, che l'Italia ha adottato nel corso degli anni, addirittura prevede tempi decisamente maggiori. maggiori. In particolare, ci sono stati dei Ministri, non Salvini, che, nella stessa identica situazione in cui si trovò l'allora Ministro dell'interno, hanno fatto attendere anche quindici giorni gli immigrati sulla nave prima di farli sbarcare, naturalmente dalla prima richiesta di porto sicuro. Nell'ottobre del 2019, al testimonianze di articoli di giornali, quando era ministro dell'interno Luciana Lamorgese, con il Governo Conte-*bis,* la nave Ocean Viking attese al largo della Sicilia dodici giorni che sono un po' più di sei - prima di far sbarcare gli immigrati. Tanto che nelle ricostruzioni, leggendo gli articoli, addirittura vi fu un *tweet* dei rappresentanti dell'Ocean Viking, che diceva: dopo più di dodici giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro. È la fine di un'odissea.

Luciana Lamorgese. La nave Geo Barents di Medici senza frontiere, con a bordo 113 naufraghi, attese ben undici giorni

per quale motivo, per sei giorni di attesa in mare un Ministro venga messo sotto processo e ci sia una richiesta di condanna, mentre per tanti altri Ministri, che hanno fatto attendere anche molti più giorni,

è più una vicenda politica. Per quale ragione? E poi noi diciamo che è una sorta di sconfitta della politica. In primo luogo, lo è perché a mandare sotto processo - così lo diciamo una volta per tutte un Ministro per decisioni politiche assunte nell'esercizio delle sue funzioni e nell'interesse nazionale è stata una parte politica. Da quella parte politica spesso e volentieri arrivano lezioni - addirittura qualcuno si erge anche a paladino del garantismo quando poi, alla conta dei fatti, si tratta della solita storia italiana, del solito garantismo italiano: garantisti con gli amici e giustizialisti con gli avversari.

che, quando non si riesce a sconfiggere un avversario con le idee o con una linea politica *(Applausi)*, si tenta di farlo attraverso le aule giudiziarie; quello che fu fatto, né più né meno, nei confronti di Silvio Berlusconi *(Applausi)*. Quindi questo cattivo costume continua ad andare avanti in questa direzione. e mi avvio a concludere - si tenta di criminalizzare dal punto di vista penale una condotta di Governo, una linea politica legittima sul tema dell'immigrazione (prima la redistribuzione e poi lo sbarco), seguita dall'allora Ministro dell'interno, ma anche dal ministro Luciana Lamorgese e dai Governi di centrosinistra e di unità nazionale che sia una limitazione della libertà di espressione politica e quindi anche democratica criminalizzare una condotta di Governo. In quarto luogo, quale segnale positivo si può dare alla popolazione quando ci si trova di fronte ad un Ministro che di fatto rispetta la volontà popolare e il programma per cui è stato eletto, ma, anziché vedersi riconosciuto il merito di questo rispetto, si ritrova sotto processo? Sono domande che noi poniamo all'Assemblea, perché oggi capita ad una parte politica, ma un domani potrebbe riguardare qualsiasi altro Ministro. Concludo dichiarando che noi siamo al fianco di Matteo Salvini e sempre lo saremo; siamo convinti

Signor Presidente, anche come Forza Italia abbiamo ritenuto di dover intervenire in ordine al processo e alla richiesta di condanna

tre ragioni che vado ad esporre. Si tratta di un processo politico innanzitutto perché l'autorizzazione a procedere appare viziata da un'evidente disparità di trattamento, motivata solo da questioni politiche. Per analogo episodio, quello che riguarda la nave Diciotti, in precedenza il Senato aveva negato l'autorizzazione a procedere. Perché una diversa valutazione su casi del tutto analoghi? Nel primo caso, durante il Governo Conte I di colore giallo-verde, il MoVimento 5 Stelle si è schierato a difesa del Ministro dell'interno e l'autorizzazione non è passata. Quando, qualche tempo dopo, si è trattato invece di votare per il caso dell'Open Arms, Salvini era passato all'opposizione e quindi è seguito il pollice verso da parte della mutata maggioranza politica, questa volta giallo-rossa. Non sussiste però, Presidente, alcuna ragionevole coerenza tra le due decisioni dell'Aula. Secondo argomento: ricorda, Presidente, la telefonata tra Luca Palamara, intercettata, e il procuratore di Viterbo Paolo Auriemma? Cosa disse il procuratore? Con argomenti giuridici, il dottor Auriemma sosteneva la legittimità dell'operato di Matteo Salvini, Matteo Salvini, cito testualmente: «Mi dispiace dover dire che non vedo veramente dove Salvini stia sbagliando. Illegittimamente si cerca di entrare in Italia e il Ministro dell'interno interviene perché questo non avvenga. Questo dal punto di vista tecnico, al di là dell'atto politico». quella che viene sindacata in sede penale è l'azione del Ministro e del Governo, una linea politica condivisibile o meno, ma una linea politica. Agli elettori il *leader* della Lega si è sempre presentato come il difensore dei confini nazionali contro l'immigrazione clandestina. I comportamenti che vengono processati a Palermo altro non sono che l'attuazione di questo suo impegno politico assunto nei confronti dei suoi elettori. Per questo, come Forza Italia giudichiamo abnorme e pericolosa la richiesta di condanna della procura palermitana ed esprimiamo a Matteo Salvini la nostra solidarietà politica ed umana.

ma se a criticare la recente sentenza della Corte di cassazione che ha annullato le condanne sul caso Ilva - peraltro una sentenza fondata su un principio assolutamente elementare giuridico, ossia l'articolo 11

Signor Presidente, sarò molto breve, perché credo che questa discussione debba essere svolta nelle sedi proprie e cioè dove viene svolta, dico da parte mia e del mio Gruppo è che per noi le valutazioni della magistratura non devono mai influire sulle valutazioni politiche, per noi l'agire del ministro Salvini è stato fallimentare dal punto di vista politico, sia come Ministro dell'interno, sia come Ministro dei trasporti. Basta chiedere a qualsiasi italiano che salga su un Frecciarossa o che cerchi un taxi alla stazione Termini. E la stessa cosa è accaduta quando era Ministro dell'interno. Sarà la magistratura a valutare se ci saranno profili penali o meno. Ma il fatto che un Ministro di un Governo in carica della nostra Repubblica abbia ignorato la legge del mare, che è una legge antichissima che regola i rapporti tra i popoli, a partire dal nostro mare Mediterraneo, che si fonda su un principio base che è quello che quando un naufrago in mare chiede aiuto, la prima cosa che si fa è tendergli una mano, penso che sia un problema che richiede una valutazione politica, soprattutto in questa sede. Sono altre le aule dove si svolgono le considerazioni giuridiche e giudiziarie e noi ci manteniamo su una valutazione puramente politica che sarebbe rimasta tale qualunque fosse stato l'orientamento del Senato sulla possibilità del ministro Salvini di essere sottoposto a giudizio e qualsiasi sarà la valutazione della Corte che lo sta valutando. Signora Presidente, ancora una volta si dimostra che la pausa estiva non fa bene agli amici della Lega, a cui in questo periodo capita spesso di prendere degli abbagli. Il senatore Romeo ha probabilmente scambiato l'Aula del Parlamento per un'aula del tribunale, perché, rispetto a quella requisitoria di difesa che ha fatto del suo *leader* Matteo Salvini, gli suggerisco caldamente di andare a deporre in tribunale. A questo correggo il collega Zanettin: in questa sede nessuno sta criticando una sentenza; siete voi che volete addirittura impedire la celebrazione di un processo. È completamente diverso. *(Applausi)*. Confesso che ho apprezzato i toni pacati che ha comunque usato il senatore Romeo, però ha detto delle cose gravi e inesatte. Criminalizzazione degli atti del ministro Salvini: se c'è qualcuno che criminalizza in maniera generalizzata le persone è proprio il ministro Salvini, ma anche gli esponenti della Lega quando chiamano qualunque migrante "clandestino", avendo già quindi emesso un verdetto di essere illegali persino sulle navi delle ONG,

nelle piazze digitali e nelle piazze popolari. Quale rispetto per gli architravi e per i pilastri della nostra Costituzione, per i tre poteri della nostra Costituzione, per l'indipendenza del potere giudiziario dimostrano Matteo Salvini e tutto il Governo, che si è sollevato in suo supporto e sostegno? Si è trattato di un uso vergognoso e in spregio delle regole democratiche ancora vigenti in questo Paese.

noi comprendiamo benissimo l'esigenza da parte del Gruppo della Lega di manifestare vicinanza e solidarietà al proprio *leader* in un momento così complicato della sua vita: sotto processo per un reato così infamante come quello del sequestro di persona.

che si colga il pretesto di questa vicenda per delegittimare la magistratura. Questo è inaccettabile ed è quello che è accaduto nei giorni scorsi. *(Applausi)*. Infatti, si è parlato di processo politico e si è messa in discussione la legittimità di un'azione giudiziaria, che si può criticare perché son criticabili certamente le singole decisioni dei giudici. non si può cogliere l'occasione, come peraltro ho sentito anche nelle parole del collega Zanettin, per tornare nuovamente a delegittimare l'intera magistratura. Non è questo che serve al Paese; al Paese non serve continuare ad alimentare questo scontro tra la politica e la magistratura. Vorrei anche al collega Romeo che non è questa la sede per fare il processo al senatore Salvini. Egli ha fatto una serie di considerazioni che verranno portate al processo, i magistrati decideranno e noi auspichiamo che il senatore Salvini esca indenne da questo processo, perché non abbiamo nessun desiderio di combattere lui e le sue idee attraverso gli strumenti

il fatto che qualunque Ministro abbia titolo e legittimità per perseguire i propri obiettivi politici lo legittimi a essere sciolto da qualunque vincolo di rispetto delle norme. *(Applausi)*. Questo è il punto su cui dobbiamo interrogarci: può il legittimo perseguimento di obiettivi politici giustificare qualunque condotta e qualunque comportamento? Può arrivare a giustificare una condotta che, in ipotesi, è quella del sequestro di persona? Questo è il punto. Non ci sono delle regole che servono anche a delimitare l'esercizio del potere? Questo è lo Stato di diritto, è il fondamento della democrazia liberale. Ritengo pertanto che noi dobbiamo difendere lo Stato di diritto e non metterlo in discussione come voi state facendo in questi giorni sul processo a Salvini. ha facoltà. MALAN *(FdI)*. Io ritengo molto appropriato l'intervento del senatore Romeo, anche perché l'attuale processo di cui stiamo parlando, il processo di Palermo, avviene perché quest'Aula, qualche tempo fa, ha dato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini.

vuol dire che un potere ha il suo ambito, nel quale ha tutta l'indipendenza che la nostra Costituzione garantisce alla magistratura, ma altrettanta indipendenza deve essere data all'Esecutivo e al Legislativo.

applicato dal Ministro, viene ritenuto però da non applicare sulla base di nobili, ma vaghi e opinabili principi principi superiori. Il principio dell'umanità è un principio che tutti condividiamo. Il punto è come si articola e come si estrinseca il principio di umanità e del rispetto dei diritti umani: attraverso le leggi, perché altrimenti è tutta valutazione arbitraria di qualcuno. qualcuno. Questo è il problema nella mancata separazione dei poteri, che si ha nel momento in cui non soltanto gli atti discrezionali, ma persino le leggi

alla forza della legge, allora abbiamo una cosa che può essere fatta, ma non da un tribunale, bensì dalla Corte costituzionale, alla quale un tribunale può arrivare, con le dovute procedure.

E non sono solo parole quando diventano un processo con una richiesta di condanna a sei anni per un Ministro dell'interno che ha svolto le sue funzioni. Pertanto credo che sia giusto che quest'Assemblea si occupi e si preoccupi del problema. Ringrazio il senatore Romeo per aver avviato questo momento di riflessione, che però è una riflessione di carattere generale. l'opposto; so che è poco verosimile, ma potrebbe accadere che un magistrato decida di inquisire un Ministro dell'interno perché non ha difeso sufficientemente i confini, perché c'è il principio della tutela della sicurezza e così via. Potrebbe succedere questo e non credo che piacerebbe a chi oggi invece ritiene che la magistratura, salvo eccezioni (come anche qui ha detto il senatore Zanettin), sia assolutamente insindacabile. Nessuno intende Nessuno intende delegittimare la magistratura verso la quale nutriamo il massimo rispetto. Ma, proprio perché ne abbiamo rispetto, riteniamo che il singolo atto del singolo magistrato possa benissimo essere criticato, anche da parte di un Ministro e anche usufruendo di uno dei mezzi di comunicazione che ci sono e che possono essere il servizio pubblico o i cento altri mezzi di informazione che ci sono. normale che il pubblico, proprio da un servizio pubblico, sia interessato a sapere quello che un Ministro ha da dire riguardo a un processo e a una richiesta di condanna così grave. voglio precisare che intervengo a titolo personale in un minuto. Naturalmente la propaganda si può sempre fare

ha la sua sede naturale all'atto dell'autorizzazione a procedere che il Senato ha concesso nei confronti del ministro Salvini. *(Applausi)*. che si rivolge nei confronti dei magistrati è in gran parte impropria. Che cosa si critica rispetto alle decisioni (che peraltro non sono state assunte possibili) della magistratura? Si critica il fatto che i magistrati, con un'interpretazione che sarà soggetta a tre gradi di giudizio, applichino la legge. Il tema vero è la sovranità della politica. La politica, cioè il Parlamento, con una decisione che io personalmente non ho avallato, ma che è stata avallata dalla maggioranza del Parlamento, dà alla magistratura la possibilità di decidere, sulla base della normativa esistente, la sorte giuridica

Parlamento. Se mi consentite, ho voluto precisare questo, al di là delle parti politiche, perché credo che l'occasione persa da parte del Parlamento sia stata in passato e certamente non possa essere recuperata oggi

Il relatore, senatore Rastrelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. il disegno di legge di iniziativa della senatrice Stefani, approvato in sede redigente, con modifiche, dalla Commissione giustizia, introduce nuove norme a tutela della classe forense in termini di legittimo impedimento. Nel corso dell'esame in Commissione, anche grazie al qualificato apporto delle opposizioni - e mi sia qui consentito ringraziare in modo particolare, per il rispettivo contributo, il senatore Bazoli e la sono stati approvati due emendamenti e due proposte di coordinamento. Il disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile il nuovo testo, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, prevede che, con provvedimento del giudice, ovvero prima della costituzione delle parti del Presidente del tribunale, sia disposta la remissione in termini del difensore che comprovi, a mezzo di idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile, ovvero comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, per assistenza a figli e familiari con disabilità o gravi patologie, ovvero per esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non consentano al difensore di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, ovvero - ancora - in caso di infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza. Il testo originario faceva riferimento semplicemente alla gravidanza, ma con modifiche approvate in Commissione, si è ritenuto di circoscrivere la rilevanza dello stato di gravidanza come causa di legittimo impedimento al solo caso in cui si determini una effettiva compromissione delle condizioni di salute della donna e si sostanzi quindi una impossibilità oggettiva di gestire il mandato. L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che disciplina il cosiddetto calendario del processo. La nuova disposizione prevede che quando il difensore non si presenti in udienza e l'assenza sia dovuta all'assoluta impossibilità a comparire per le circostanze già indicate, il giudice debba disporre il rinvio a nuova udienza. Questo naturalmente purché le circostanze siano comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza ovvero, secondo la modifica introdotta all'originario disegno di legge dalla Commissione, comunicata alla cancelleria del giudice che procede, anche a mezzo PEC, nei medesimi termini. Da ultimo, l'articolo 3, non modificato dalla Commissione, interviene sul comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina il legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del quinto comma nella formulazione vigente il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore quando risulti che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato. Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che possono costituire cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore. Il disegno di legge, Presidente, va pertanto nella direzione di un rafforzamento delle garanzie del difensore, di un deciso contrasto a comportamenti, prassi e consuetudini, che costituiscono peraltro una vera e propria discriminazione nei confronti dell'avvocatura perché comportano una evidente disparità di trattamento tra giudici e avvocati difensori. Con il provvedimento si vuole infatti evitare che la valutazione di taluni impedimenti sia lasciata alla libera interpretazione, quando non anche all'arbitrio, di un collegio giudicante con decisioni che comportano spesso il rischio di decadenza da termini processuali perentori. Il diritto di difesa dei cittadini deve infatti essere sempre garantito ciò può essere fatto anche prevedendo espressamente, come causa di legittimo impedimento, caso fortuito, forza maggiore o altri eventi che l'esperienza delle aule di giustizia segnala come necessari per determinare un quadro normativo che sia in grado di coniugare ragionevolmente il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria con la tutela dei difensori in presenza di situazioni particolarmente gravi. Ciò significa, come è evidente, operare sempre per la salvaguardia della posizione processuale dei loro assistiti e quindi per la tutela dei cittadini.

sono "animali" rarissimi che vediamo pascolare in quest'Aula, quindi, quando un disegno di legge d'iniziativa parlamentare arriva alla nostra approvazione, la Camera e il Senato dovrebbero celebrarlo. È un disegno di legge che evidentemente va a riempire un vuoto va a riempire un vuoto essenziale. Abbiamo ascoltato la relazione del relatore senatore Rastrelli, che ci ha spiegato tecnicamente di cosa stiamo parlando;

che sarebbe doveroso e lodevole - lo sforzo di realizzare quel principio per il quale accusa e difesa devono essere uguali e pari davanti al giudice terzo. È il principio che ispira il

Ma c'è anche - ed è il profilo che mi preoccupa maggiormente - un racconto dell'azione penale che acquisisce, di giorno in giorno, di mese in mese, sempre più un aspetto di tipo quasi vendicativo, come a dire «giustizia è fatta», di esemplarità della pena. Un processo penale viene descritto sempre con l'imputato che è, di fatto, il cattivo del film, mentre i buoni sono tutti dall'altra parte, e giustizia è fatta quando l'imputato viene condannato, possibilmente a una pena esemplare, con buona pace dei principi costituzionali della presunzione di innocenza, per esempio, per cui ogni imputato è innocente fino a sentenza definitiva. Anche il racconto giornalistico dei processi è, nella stragrande maggioranza dei casi, ispirato a principi giustizialisti, al facciamo vedere la giustizia nella sua implacabilità, nella sua forza che schiaccia chi ha sbagliato. Io penso che questo non sia il processo penale che avevano in mente i nostri Costituenti e non è il processo penale come dovrebbe essere in un Paese maturo dal punto di vista della sua civiltà giuridica, come l'Italia, la patria di Beccaria, la culla del diritto. Pertanto, anche disegni di legge piccoli come questo ci aiutano a ristabilire una realtà una realtà del processo penale che si inserisce meglio dentro quei parametri che descrivono il processo penale per la nostra comunità nazionale, per il nostro Paese, per la nostra Costituzione. La giustizia, per come viene rappresentata, ha in mano una spada ma anche una bilancia ed è bendata perché non deve guardare in faccia a nessuno, ma deve farlo con severità ed equilibrio. Allora andiamo a regolamentare dei principi che consentano di dirci se l'avvocato può non esserci, salvo naturalmente che non ci siano più avvocati a difendere l'imputato e salvo che non si tratti di ragioni non fondate. Però, se l'avvocato o l'avvocata - perché per fortuna nelle nostre aule giudiziarie, tanto tra la magistratura che nelle professioni forensi ci sono molte donne, spesso nella nostra società, ahimè, è ancora molto collegato a compiti di assistenza familiare - hanno impedimenti che vanno ad incidere nella dinamica processuale, è giusto che la nostra Costituzione, quella dell'articolo 3,

il quale o la quale non veniva messo o messa in condizione di poter opporre una circostanza familiare, come quelle che bene ha elencato il senatore Rastrelli come elemento di fermo della procedura. Poi l'ingiustizia, come sempre succede con le ingiustizie, signora Presidente, va sempre a colpire i più deboli, anche quando l'apparente vittima di un'ingiustizia è un po' più forte, c'è sempre qualcuno nella catena che che ne subisce gli effetti finali. In questo caso è l'imputato, perché l'impossibilità di esercitare il proprio mandato di difensore si tramuta alla fine, nell'anello più debole, in una penalità per l'imputato che deve far fronte alla legge senza l'assistenza legale necessaria. Allora, è un piccolo disegno di legge che afferma un grande principio.

il testo su cui oggi siamo chiamati a votare ha il fine di rimuovere la disparità di trattamento che esiste oggi tra giudici e avvocati nell'esercizio delle loro funzioni. Mentre per i magistrati è possibile, infatti, rinviare anche più volte le udienze per impedimenti personali, per i legali spesso persino una situazione familiare improvvisa e fortemente preoccupante non giustificava fino ad ora la richiesta di rinvio. Il rischio denunciato più volte dalla categoria forense è quello di una compromissione del principio di indipendenza ed autonomia nell'esercizio del diritto di difesa. Più volte notizie di stampa hanno riportato il caso di avvocati ai quali è stato di fatto negato il diritto di un rinvio per assistere il proprio figlio, senza parlare di quelli in cui il difensore stesso, per ragioni di salute personali, è incorso in decadenze processuali non rimediabili. Questo disegno di legge colma quindi un vuoto normativo del processo civile, introducendo la possibilità per il difensore di venire rimesso in termini quando dimostra, con idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per cause a lui non imputabili, o comunque derivanti da fatto fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o, per esempio, gravidanza; per assistenza a figli, familiari con disabilità o grave patologia; esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o scolare che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. Inoltre, è consentito il rinvio dell'udienza se l'avvocato non può comparire per le medesime ragioni. Inoltre, anche nel processo penale, il legittimo impedimento del difensore (articolo 420-*ter*, comma 5, del codice di procedura penale) verrebbe esteso ai casi di malattia della prole o dei familiari. Noi riteniamo quindi che si tratti di una norma di civiltà che deve essere riconosciuta quale diritto per gli avvocati e le avvocate, spesso nell'esercizio delle loro funzioni da problemi di salute propri o dei familiari, o da cause di forza maggiore. Di conseguenza, annuncio il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra.

è un disegno di legge molto opportuno, che va a colmare una lacuna dell'ordinamento. Fino ad oggi, infatti, quello che era il legittimo impedimento del difensore, sia nel processo civile che nel processo penale, non era normato in modo adeguato le cause di forza maggiore, piuttosto che gli impedimenti legati alla famiglia, piuttosto che alle malattie, non costituivano motivo obbligatorio per il rinvio. L'*occasio legis*, come poi spiegherà meglio la collega Stefani, nasce proprio da un evento personale che l'ha interessata, che ha riguardato per certi versi l'intero Foro vicentino, al quale io pure appartengo. Da questo episodio di vita concreta, di vita processuale concreta, che, nel caso di specie, come spiegherà meglio lei, è stato risolto, ma attraverso la cortesia di colleghi e la comprensione dei magistrati, si è messo a fuoco un problema serio, un problema concreto, un problema reale, che riguarda appunto la possibilità che avvocati che si trovano in condizioni di difficoltà improvvise, imprevedibili, per cause di forza maggiore o collegate a patologie mediche piuttosto che alla gravidanza, riescano a risolvere la questione. Ciò perché, invece, episodi, anche questi di vita concreta, di vita processuale concreta, all'interno delle aule di giustizia, hanno dimostrato come collegi piuttosto che magistrati troppo intransigenti a volte non erano nelle condizioni o non volevano risolvere problemi di questo tipo. Da questo punto di vista, si va a colmare un vuoto normativo, che sussisteva e che non era sanabile, perché la possibilità di avere i collegi congiunti, cioè due avvocati che

evidenziato dalla collega è assolutamente un tema importante. Come ha detto prima il collega Scalfarotto, questo è un disegno di legge molto puntuale, che riguarda una fattispecie specifica, ma che illustra un tema generale, cioè la tutela del cittadino, la tutela dell'avvocato di fronte a un magistrato che, come è stato ricordato anche poc'anzi, viceversa ha la possibilità di disporre rinvii anche *ad nutum*, senza particolari giustificazioni. Ciò era inspiegabile nell'ottica della parità fra fra difesa e accusa, che è uno dei cardini del Dna di Forza Italia, tant'è che lo decliniamo anche nella riforma della separazione delle carriere. È un punto assolutamente qualificante, un principio assolutamente condiviso, condivisibile e legittimo. Quindi, da questo punto di vista, non posso che confermare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. colleghe, partendo dal presupposto che esercito la professione forense da ventotto anni, e che quindi non vi sono né preconcetti né ritrosie a muovere i miei ragionamenti, il mio sarà un discorso prima di tutto tecnico e successivamente politico. Dal punto di vista tecnico, il disegno di legge muove da un intento che è sicuramente degno di nota. Ribadisco che, di mestiere, sono *in primis* un avvocato e poi, chiaramente, un politico. Il legittimo impedimento è un istituto a tutela della libera professione e concerne l'incolpevole situazione di fatto che, avendo natura assoluta e attuale, non lascia al soggetto alcuna possibilità di presentarsi in udienza, ovvero di delegare le funzioni del proprio mandato. mandato. Qui non sto a raccontare le mie esperienze personali in ventott'anni, ma io ho avuto due gravidanze, con una serie di difficoltà, anche durante l'esercizio della professione. Purtroppo, ho avuto un figlio che non è stato benissimo. Quindi, l'argomento mi tocca particolarmente ed è certamente una questione degna delle migliori attenzioni. Il disegno di legge centra in generale il problema, quale questione naturale da affrontare, ma allo stesso tempo non sembra esente da sollevare interrogativi, che più volte ho evidenziato anche in Commissione. Vengono disciplinate tre diverse tipologie di situazioni nelle quali il legittimo impedimento può palesarsi. Relativamente al settore del diritto civile, l'avvocato può invocare l'istituto in parola nei casi, tassativamente elencati, di mancata presentazione all'udienza ovvero nei casi di mancato compimento di un atto nei termini perentori previsti, al decorrere dei quali derivi una decadenza; nel penale, invece, si può invocare l'istituto nell'assoluta impossibilità a comparire in udienza. Ci troviamo di fronte a interessi ugualmente meritevoli di tutela: la salvaguardia del diritto di difesa e il giusto processo e la sua ragionevole durata. Il disegno di legge avrebbe meritato un supplemento di riflessione. Fino all'ultimo, come Gruppo eravamo indecisi se chiedere la rimessione in sede referente del provvedimento, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, perché il disegno di legge rappresenta un buon punto di partenza, ma non è esente da difetti, in quanto sicuramente perfettibile. Tutto l'arco parlamentare ne sono sicura - ha il pieno interesse nel far sì che si abbia una compiuta e ragionevole normativa relativamente al legittimo impedimento (ci sono infatti avvocati in ogni Gruppo politico). Abbiamo pensato alla sede referente proprio per far sì che la Camera non si trovasse nelle condizioni di dover modificare il testo, ovvero di approvarne uno imperfetto. Volendo, siamo ancora in tempo a farlo, qualora vi sia una volontà precisa da parte di tutta l'Assemblea di modificare il testo rendendo maggiormente tassative le ipotesi ivi previste. Il testo così formulato si presta, da un lato, a comportamenti opportunistici da parte dell'avvocato e, dall'altro, espone il professionista a una grande incertezza dovuta all'arbitrio del giudice nel valutare la richiesta. Questo lo dico come civilista. Infatti, per come è stato tipizzato il legittimo impedimento in relazione alla richiesta di rimessione in termini, fa sì che l'avvocato di controparte possa strumentalmente far scadere il termine di deposito delle memorie e beneficiare del deposito entro i termini dell'altra parte, e contestualmente usufruire della richiesta di remissione in termini per il legittimo impedimento, anche in ragione della mera assistenza dei figli. In soldoni, alla fine andrebbe a depositare una sorta di memoria di replica. A questo punto pongo una domanda all'Assemblea: quale potrebbe essere una motivazione tale da far scaturire il legittimo impedimento nei casi di assistenza ai figli? L'adempimento dell'obbligo scolastico mediante l'assolvimento del dovere di accompagnare i bambini a scuola potrebbe essere un motivo tale da far accoglie una richiesta di legittimo impedimento? Di converso, quali potrebbero essere le ragioni di accoglimento da parte del giudice della richiesta di legittimo impedimento relativamente alle esigenze improrogabili e di cura della prole in età scolare tale da non consentire al professionista di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato? Per come è scritta la norma, o non verrà mai concesso il legittimo impedimento e quindi questo disegno di legge risulterà assolutamente inutile, oppure aumenteranno a dismisura i casi in cui verrà concesso, con conseguente paralisi dell'attività giurisdizionale. La certezza del diritto nonché la ragionevole durata dei processi sarebbero inficiate da un'interpretazione della norma in tal guisa. Nel caso invece di cui all'articolo 2, ovvero quello relativo alla richiesta di rinvio di udienza, una lettura costituzionalmente orientata lo vedrebbe rapportato al principio del giusto processo, ma solo qualora il rinvio del termine dell'evento impeditivo fosse breve tale da garantire la ragionevole durata del processo.

Quando si ragiona di legittimo impedimento, signor Presidente, si deve pensare sia agli effetti in capo alla parte attrice, sia alla parte convenuta. Pensiamo infatti al creditore che non riesce a soddisfare la propria pretesa creditoria oltre ogni ragionevole dubbio di diritto. La tutela del legittimo impedimento deve essere quindi bilanciata con il diritto di difesa della controparte. C'è un evidente problema di bilanciamento, di interessi in un giudizio: in questo caso ho fatto l'esempio del creditore e del debitore. Come MoVimento 5 Stelle avevamo predisposto molteplici proposte: alcune sono state assorbite da emendamenti approvati; altre sono confluite in ordini del giorno accolti dalla Commissione; altre ancora, purtroppo, non sono state prese in considerazione e questa circostanza dispiace molto. C'è stato un gran lavoro ma - lo ripeto - potevamo fare molto di più. Veniamo ora alla parte politica. Il provvedimento che interessa l'Assemblea è il classico esempio di disegno di legge che poteva essere approvato all'unanimità. In Commissione ci siamo astenuti, anche se ne condividiamo gli obiettivi. Siamo ancora in tempo per fare un lavoro unitario. Nessuna legge nasce perfetta, figuriamoci un disegno di legge. Queste le parole della relatrice durante le audizioni, parole che condivido appieno. Su questo disegno di legge si potrebbe lavorare a quattro mani. La norma necessita di un intervento: lo sapete voi come lo sappiamo noi. Non chiederemo la referente, anche se il disegno di legge necessiterebbe di questa trasformazione. Siamo certi che lo farete voi affinché possa essere riaperto il termine di presentazione degli emendamenti. Nel frattempo, non potendo votare contro il disegno di legge perché consideriamo improcrastinabile un intervento legislativo sulla materia, ci asterremo dal votare, viste le numerose suesposte criticità che necessitano di un'accorta revisione del testo. *(Applausi)*.

ricordare, *in primis*, che la Costituzione sancisce che la difesa è un diritto inviolabile. La difesa è in parte a carico e di responsabilità dell'avvocato.

non riconoscendosi l'importanza fondamentale di tale figura all'interno di un processo e nel sistema stesso della giustizia. La giustizia necessita chiaramente dei magistrati, degli apparati, dei tribunali, dei Ministeri, ma soprattutto degli avvocati.

ero stata colpita da un'emorragia cerebrale che mi ha portata immediatamente in una situazione di coma che è durata quasi una settimana. Chiaramente non avevo la possibilità né di delegare, né di indicare un sostituto, né di avvisare il cliente che non ero più in grado di rispettare un termine o di presenziare un'udienza (questo accade in particolare nel settore civile, l'ambito nel quale esercito). Questo *vulnus* è stato per certi versi sanato nel caso che mi ha riguardato dalla cortesia di colleghi di controparte, dalla cortesia di magistrati, dalla cortesia anche di colleghi che si sono presentati al mio posto, nella stessa udienza, chiedendo impropriamente, pur non avendo una delega, il rinvio. non può essere che un sistema funzioni e che i diritti degli assistiti siano garantiti a seconda che vi sia un'eleganza, una cortesia da parte di colleghi o di magistrati.

questo sistema sia bilanciato e che il dibattito che c'è stato in Commissione sia stato molto fruttuoso, anche perché è stato coadiuvato e arricchito

giustificare anche un rinvio di un'udienza o una rimessione in termini, è importante. Nonostante questo abbiamo qualche dubbio su come le norme sono state formulate (dubbi che abbiamo espresso durante l'istruttoria)

Non possiamo dire, come è sembrato di intendere da questo dibattito, che non ci sono norme che tutelano il difensore

in discussione cerca di specificare e di dettagliare i motivi che possono giustificare il legittimo impedimento. Bisogna tuttavia ricordare che su quelle norme c'è già una montagna di giurisprudenza.

interpretano male o applicano male le norme, non seguendo la giurisprudenza consolidata, ma sono abbastanza sporadici. Ci sono le norme deontologiche che riguardano l'avvocatura, perché ovviamente c'è anche una responsabilità degli avvocati nel consentire o non consentire, per esempio, un rinvio di udienza. Ho sentito parlare di parità tra accusa e difesa e di riequilibrio dei poteri tra giudici e avvocati. Ma, colleghi, qui stiamo parlando soprattutto di processo civile: due articoli su tre riguardano il processo civile, che è un processo tra parti private,

il rapporto è tra parti private. Quindi il riequilibrio tra accusa e difesa, tra giudice e avvocati dove lo vedete? Cosa c'entra con questo provvedimento? Questo è il punto. Il modo con cui sono stati dettagliati i motivi che giustificano la rimessione in termini e il rinvio di udienza nel processo civile

per consentire di mettere al riparo quella norma dal rischio di comportamenti opportunistici, che nel processo civile sono ben ben possibili. Nel processo civile, tendenzialmente e tradizionalmente, c'è una parte che chiede e una parte che deve dare, c'è un creditore e un debitore. Il debitore tendenzialmente, finché può, cerca di non pagare e quindi cerca di dilazionare i tempi per arrivare a una decisione. Se noi offriamo degli strumenti, che possono essere utilizzati male, a qualcuno che ne approfitta, non facciamo un servizio alla giustizia, ma rischiamo di mettere qualche mettere qualche granello di sabbia in più nel funzionamento dei nostri processi nei nostri tribunali. Quello che abbiamo cercato di fare in Commissione è offrire delle occasioni e delle opportunità di miglioramento del testo. Siamo

questo provvedimento non ha una natura politica, ma ha una natura prettamente tecnica, quindi non ci sono ragioni di natura politica per le quali uno può essere a favore o contro. Ci sono ragioni di natura tecnica e io mi auguro che, nel passaggio che si farà alla Camera, ci sia la disponibilità, per una volta, a non continuare a consolidare questa sorta di monocameralismo di fatto, per cui

Pur condividendo in linea di principio gli obiettivi che sono stati assegnati a questo disegno di legge, pensiamo che si sarebbe potuto fare un lavoro molto più accurato e molto più efficace.

È innegabile che sono molteplici i casi in cui il legittimo impedimento dei difensori non viene riconosciuto dai giudici sia nel civile, che nel penale. Molte istanze di rinvio dovute al legittimo impedimento non vengono accettate con la motivazione che ci si può far sostituire dal collega di studio, che però non ha la delega nel procedimento in corso. È capitato pure a me, anche nella mia funzione di parlamentare, chiedendo un rinvio da avvocato. Come ha detto la senatrice Stefani, capita anche in casi gravi ed estremi. Sempre per non parlare di altri: alla mamma di mio figlio è stato negato un rinvio nonostante fosse in gravidanza a rischio, perché poteva farsi sostituire da una collega. Nel caso in cui il rinvio non venga concesso, l'avvocato fa una figuraccia, ma chi paga le conseguenze del mancato rinvio e, quindi, del processo che si fa in assenza del legale che è stato individuato come fiduciario da parte della persona patrocinata? Ne paga le conseguenze il difeso, il cliente, ossia colui che si affida

che da tutelare sia il cittadino, ancor prima delle esigenze dell'avvocato. Crediamo che questo provvedimento garantisca all'avvocato di vedersi tutelato in determinati casi particolari che sono ben enunciati nel provvedimento, affinché egli possa meglio tutelare il cittadino che si è affidato alle sue cure. Cosa si può fare di meglio? Tutto è migliorabile e certamente non sosteniamo che il provvedimento sia perfetto. se voi tutti e noi tutti condividiamo che vi sia la necessità di un intervento urgente - prima si fa, meglio è (concordo anche su questo) - perché non votare intanto il provvedimento? Perché negare che, a oggi, il legittimo impedimento, così come concepito, non funziona né nel procedimento civile, né in quello penale? Perché negare che il cittadino ha il diritto di vedersi difeso dall'avvocato che ha scelto? Perché l'avvocato che è stato scelto deve, senza motivo, delegare a un altro collega o non collega di studio il dovere di difendere il cittadino che lo paga e che ha riposto in lui la sua fiducia? Poi, come giustamente è stato detto, esiste la deontologia professionale che impone di andare a vedere quali sono i casi in cui l'avvocato, con intento dilatorio, finge un malessere o un legittimo impedimento. È però l'Ordine degli avvocati che deve andare a vedere, su denuncia di eventuali colleghi, che cosa ha fatto l'avvocato, oppure c'è anche la possibilità che il giudice disponga la visita a domicilio per verificare se l'avvocato è veramente malato o ha un legittimo impedimento.

Penso che nessuno di noi abbia mai fatto un esposto per questo. Come capita ai giudici e ai magistrati, può capitare anche ai cittadini, e quindi agli avvocati, di avere un legittimo impedimento, un malore improvviso, una causa di forza maggiore. In questo caso dobbiamo sempre difendere la persona che a quell'avvocato si è affidata. Ancor di più nell'articolo 1, che concerne le decadenze; se per un legittimo impedimento di un avvocato il cliente incappa in una decadenza non più sanabile, perde la causa, è impossibile difenderlo, non si può più fare appello in caso di condanna penale? È corretto questo? Noi pensiamo che sia corretto tutelare quel cittadino

il provvedimento solo perché ha due articoli su tre riguardanti la procedura civile non coinvolga anche il procedimento penale; lo fa bene e ampiamente nell'articolo 3.

e dando ai loro - nostri - clienti la possibilità di non aver paura che il legittimo impedimento del proprio difensore non venga accettato. Per questo motivo, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento

Il relatore, senatore Paganella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 925, di cui la 7a Commissione permanente ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 17 luglio. Il disegno di legge, a prima firma del presidente della 7a Commissione, senatore Roberto Marti, reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale del formatore. Esso si compone di quattro articoli. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Repubblica riconosce il giorno 14 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale del formatore. La data scelta, come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, ricade nel periodo dell'anno in cui prende avvio prende avvio l'anno scolastico e della formazione professionale. Al comma 2 si precisa che non si tratta di una ricorrenza festiva. Le iniziative celebrative che mirano a promuovere la conoscenza della centralità dell'attività dei docenti e dei formatori sono disciplinate dagli articoli 2 e L'articolo 2 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali hanno la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, eventualmente anche con il coinvolgimento delle associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori. L'articolo 3, a seguito di una modifica, peraltro unica, introdotta in sede redigente, dispone che le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale nonché gli istituti tecnologici superiori possano, nell'ambito della loro autonomia, promuovere attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere. L'articolo 4 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria. Come precisa la relazione illustrativa, la finalità del provvedimento è quella di dedicare una giornata nazionale di analisi, studio, riflessione, discussione e proposta a docenti e formatori, per creare un'osmosi di esperienze da valorizzare in Italia e nel mondo, e di sottolineare il loro ruolo nel campo della cultura, dell'istruzione, della formazione e della solidarietà, che risulta centrale anche per la diffusione dei principi democratici. La proposta legislativa si inquadra peraltro nell'ambito della promozione dell'importanza delle professioni di docente e formatore messe in atto dal Consiglio dell'Unione europea, con proprie iniziative diffusamente richiamate nella relazione illustrativa.

Signora Presidente, sarebbe facile fare dell'ironia sull'ennesima giornata celebrativa, ma il Gruppo per le Autonomie voterà a favore di questo provvedimento, perché è giusto e doveroso celebrare la funzione sociale dei formatori, degli insegnanti, degli educatori, di chi opera per migliorare il lavoro delle imprese, della pubblica amministrazione, di chi aiuta quelli che hanno perso il lavoro a rientrare nel mondo dell'occupazione. Ognuno nella vita ha avuto un insegnante o un educatore che ne ha segnato il percorso e chissà come sarebbero andate le cose se non l'avesse mai incontrato. Chi forma agli altri alla vita o al lavoro ha una grande responsabilità; è la promessa che l'impegno e il sacrificio di oggi verranno riconosciuti da una società in cui ciascuno troverà il proprio spazio e la propria strada. Ma la domanda che dobbiamo porci, Presidente, è cosa significa formare in questo nostro mondo globalizzato e iperconnesso, della crisi democratica e delle *fake news*, un mondo che, con l'intelligenza artificiale, si avvia al più grande sconvolgimento dei modelli produttivi, degli assetti sociali e dei processi economici dai tempi della rivoluzione industriale. Formare significa innanzitutto sapere, nell'accezione data da don Lorenzo Milani: «La scuola - diceva don Milani - è l'arte delicata di condurre i ragazzi sul filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della legalità (…), dall'altro la volontà di leggi migliori cioè di senso politico». Formare significa quindi costruire una cittadinanza matura e consapevole dei propri diritti e doveri, che partecipa attivamente e con cognizione di causa al processo democratico, ma formare in questa nostra società significa anche accompagnare i processi di cambiamento. Dobbiamo cioè uscire dall'idea della formazione come addestramento per migliorare le abilità individuali per andare incontro a un'idea della formazione come pilastro strategico nelle politiche per l'innovazione e la competitività. È quindi una formazione che sempre più diventa un tema trasversale, che cioè non si limita solo agli anni della scuola e dell'università, ma accompagna il cittadino e il lavoratore per tutte le fasi della sua vita. È un vero e proprio salto di paradigma, anche rispetto alla figura stessa del formatore: non più o non solo una persona che trasmette un pacchetto di competenze, ma che anticipa i tempi, che capisce quali saranno i bisogni futuri, che è in grado di contestualizzarli nella cornice della costante trasformazione tecnologica. È chiaro che questa nuova visione chiama a una riflessione sulla natura del sistema universitario e della ricerca, sulla necessità di politiche di sviluppo industriale pensate attorno all'idea della formazione permanente, ed è altrettanto chiaro che un sistema che punta finalmente sul sapere non mortifica chi svolge queste professioni e penso innanzitutto agli stipendi, tra i più bassi d'Europa, dei nostri maestri e insegnanti. Per concludere, signora Presidente, noi pensiamo che sia questo il vero terreno di gioco, al di là dei riconoscimenti, delle giornate e delle celebrazioni: formazione come cultura della cittadinanza, formazione come cultura dell'innovazione, formazione come restituzione della dignità sociale a chi, dalle scuole al terzo settore, svolge ogni giorno questo lavoro. È con questi auspici che ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento.

ancora una volta ci troviamo in quest'Aula con provvedimenti che vogliono solo e semplicemente celebrare una giornata nazionale. Ormai possiamo dire una giornata nazionale non si nega più a nessuno, salvo che ormai le giornate, anche quelle nazionali, prima o poi si esauriranno, perché il calendario dei giorni è quello che conosciamo. Al di là delle battute, su cui invece c'è poco da ironizzare, il tema vero rimane tutto fermo lì: è quello della scuola, dell'istruzione, della formazione. Proprio giovedì scorso il nostro Gruppo Italia Viva ha presentato un *question time*, su cui il ministro Valditara non ha dato alcuna risposta o certezza, sulla questione ormai eterna del precariato. però una differenza: se questo problema ce lo portiamo da tantissimi anni e sicuramente non è soltanto di questo Governo, mai come quest'anno (2024-2025) daremo un anno scolastico di incertezza ai nostri studenti, alle nostre studentesse e alle famiglie italiane, perché si è raggiunto il numero *record* di supplenti e di precari, non solo come insegnanti, ma anche del personale amministrativo della scuola. Questo per dire che, se non mettiamo le risorse necessarie sulla scuola, non ne usciremo neanche con questo Governo, perché ancora una volta - e lo sappiamo dopo il Covid in modo particolare - ai nostri insegnanti, che sono gli educatori dei nostri figli, abbiamo delegato ancora di più una situazione complessa e difficile, dovuta anche al disagio giovanile e psicologico dei nostri ragazzi dopo aver affrontato due anni di pandemia.

su scala europea. Ormai abbiamo raggiunto anche questo *record* negativo: sono gli insegnanti che hanno gli stipendi più bassi in assoluto al mondo, perché non abbiamo una riforma organica del sistema scolastico e del modo in cui vogliamo incidere sulle scelte di un futuro che si presenta sempre più incerto. Al di là della Giornata nazionale del formatore, formatore, che va bene per ricordare il loro lavoro - credo che tutti possiamo essere d'accordo nel ringraziare tutti gli insegnanti, gli educatori e i formatori che ogni giorno svolgono, da eroi, un lavoro straordinario e difficile sul territorio nazionale - per tutte queste ragioni, vorremmo vedere però qualcosa di concreto e non solo la Giornata nazionale. Penso, ovviamente, alla manovra finanziaria ormai alle porte, quale vorremmo che ci fossero investimenti su tutto quello che riguarda il *welfare*, la vita quotidiana dei nostri cittadini e in modo particolare delle nuove generazioni.

della nostra società, in modo particolare scuola, *welfare*, sanità e lavoro, che sono i temi che riguardano i nostri cittadini. Per tutte queste ragioni, signora Presidente e Governo, siamo quindi costretti ad esprimere un voto di astensione, anche se speriamo che prima o poi - e su questo il Gruppo Italia Viva

del ministro Valditara sono quelle che abbiamo sentito giovedì scorso in risposta al nostro *question time,* c'è poco da sperare. *(Applausi)*. Signor Presidente, inizio subito col dire che riempire il calendario di giornate dedicate a qualcosa o a qualcuno, come questa maggioranza sta incentivando continuamente, non risolve nessun problema; anzi, credo che sia un elemento di grande retorica.

che è quello del ruolo, del valore e quindi anche della sicurezza che il formatore deve avere nella società. Non si tratta di un fatto puramente evocativo e di un momento puramente simbolico, ma deve essere un fatto concreto.

Signor Presidente, il disegno di legge di iniziativa parlamentare intende celebrare, attraverso una Giornata ad essa dedicata, la figura del formatore. Ho sentito la senatrice Sbrollini dire

ma non solo loro, posto che ormai si va verso un mondo del lavoro in cui la cosiddetta formazione continua rappresenta il fulcro per poter passare da un lavoro a un altro e spesso da un settore all'altro. Le statistiche, come quelle elaborate dalle camere di commercio italiane, ci dicono quanto pesi la carenza di talune figure professionali in Italia: centinaia di richieste di lavoro rimangono inevase, con nocumento per il sistema delle imprese italiane. Si va verso un sistema educativo e formativo sempre più qualificato e, allo stesso tempo, verso specializzazioni che si sommano alle precedenti. Il miraggio del titolo di studio unico e del posto di lavoro unico coinvolge sempre meno persone; anche chi ha già un diploma si trova a doverne prendere un altro o un'altra specializzazione, in un mondo in cui l'innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale nel far finire oppure nel creare posti di lavoro. Anche chi si occupa di formazione deve inseguire gli sviluppi di un mondo del lavoro sempre in evoluzione e adattare la sua preparazione per trasmetterla ai propri discenti. Ecco quindi che celebrare la Giornata del formatore significa celebrare un mondo dell'educazione, della scuola, della solidarietà e del lavoro in continua hevoluzione, dove si tende a conservare i vecchi mestieri e a seguire quelli nuovi. l'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale oggi: rappresenta la rivoluzione industriale di questo secolo, ma anch'essa, in un futuro che comunque è dominato dalla volontà dell'uomo, deve essere considerata una forma di supporto e aiuto, così come le macchine sostituirono taluni lavori manuali e ripetitivi e le catene di montaggio, l'intelligenza artificiale sostituirà qualche lavoro dei cosiddetti colletti bianchi. Oggi per tutti è ormai possibile trovare lezioni *on line* su quasi tutto lo scibile umano. Crediamo però che risulti difficile vedere sostituito il ruolo fondamentale del formatore, specialmente ora che la griglia delle materie offerte dalla formazione professionale si è ampliata, perché alla base della formazione sta proprio il rapporto umano. Il formatore è colui il quale, con il proprio carisma e con la passione con cui insegna, rende la lezione un evento da seguire, da non perdere. Il formatore possiede quel cuore che è ancora fondamentale a trasmettere l'amore per la materia insegnata ai propri alunni, un cuore che invece non possiedono le macchine o i *software* dotati di grande intelligenza. Il formatore è colui al quale ci si rivolge al termine della lezione per avere chiarimenti e stabilire quell'indispensabile contatto umano tra docente e discente.

potuto essere aggiunta quella degli educatori, come aveva proposto un emendamento dei colleghi del PD. Detto questo, a nostro avviso la scuola ha bisogno di risorse e di trovare una soluzione per il precariato, quindi riteniamo che questa Giornata del formatore sia semplicemente un modo per riempire la Commissione di provvedimenti poco utili. Certamente ci asteniamo perché non vogliamo andare contro un'iniziativa che può sottolineare l'importanza del formatore. Le risorse ci sembrano veramente ridicole, ma soprattutto, con questa dichiarazione di voto e importante dal punto di vista scolastico, vorrei che fosse lasciato agli atti che per il MoVimento 5 Stelle, finché alla scuola non vengono date risorse - ricordo che con questo Governo vengono dati 7 euro a scuola per l'educazione civica

Talvolta serve il ricordo, talvolta serve la giornata, ma talvolta serve lavorare su provvedimenti che possano riempire realmente di contenuti non solo economici, ma anche strutturali il mondo che abbiamo davanti. Credo che sia preciso per alcuni aspetti e impreciso per altri parlare di riempire di contenuti economici e strutturali legislativi il mondo della scuola. Questo Governo la nostra Commissione stanno ormai lavorando da ventidue mesi su tanti provvedimenti importanti, sicuramente in un mondo complesso e complicatissimo, solo perché abbiamo la premura

Il Consiglio dell'Unione europea il 9 giugno 2020, nelle sue conclusioni sui docenti e formatori del futuro, pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ricorda come l'istruzione e la formazione, oltre che a plasmare l'umanità e a promuovere la trasformazione sia delle persone sia della società, siano importanti per la partecipazione di tutti i cittadini, a livello sociale, economico, demografico e culturale, alla crescita, allo sviluppo sostenibile, alla coesione sociale e alla prosperità in seno all'Unione. Un'istruzione e una formazione di qualità, pertinenti, inclusive ed eque infatti non offrono ai cittadini solo conoscenze, capacità e competenze in linea con gli sviluppi attuali e futuri, ma ne plasmano anche gli atteggiamenti, i valori ed i comportamenti, consentendo loro di progredire. In un contesto di costanti cambiamenti sociali, demografici, culturali, economici, scientifici, ambientali e tecnologici, il mondo dell'istruzione e della formazione si sta evolvendo, come abbiamo detto prima, e la Giornata del formatore sarà un'occasione che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni potranno sfruttare, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, per organizzare iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale del formatore. Le associazioni interessate potranno avere un ruolo di rilievo per sollecitare e coordinare questi eventi, affinché ci sia un ritorno effettivo sull'intera collettività. Ovviamente, anche le scuole di ogni ordine e grado potranno scegliere di utilizzare questa Giornata per rinsaldare il rapporto docente-discente e far riflettere così i nostri ragazzi sull'importanza di avere maestri di vita, prima ancora che di ciascuna disciplina di studio. Questo Governo ha riportato la scuola e l'università al centro dell'agenda politica. Il nostro Paese vanta una tradizione millenaria nella formazione, riconosciuta oltre i confini europei, come confermano i *ranking* delle migliori università del mondo. Certo, Certo, siamo consapevoli che ci siano tanti i fattori su cui c'è un grande margine di miglioramento e grazie ai fondi del PNRR e agli investimenti garantiti dal Ministero stiamo colmando anche questo grande divario. Mi auguro quindi vivamente che questa proposta possa incontrare, sia pur con qualche eccezione e con qualche astensione, la massima convergenza, perché è evidente che l'importanza della formazione stia a cuore a tutti noi, senza distinzione di appartenenza politica. *(Applausi)*.

Ringrazio altresì il relatore, senatore Paganella. Tuttavia, vorrei subito dire in premessa che il disegno di legge in esame può certamente rappresentare un momento importante per tutte e tutti coloro che lavorano nell'ambito della formazione. Il Gruppo Partito Democratico queste ragioni le ha riconosciute anche nel lavoro della Commissione, lavorando e proponendo emendamenti. Istituire quindi una giornata, il 14 settembre, pensata per promuovere la professione ed il lavoro che i formatori svolgono ogni giorno rappresenta una proposta certamente condivisibile, ma purtroppo trovo inutile girare intorno al fatto che il presente disegno di legge manca degli elementi fondamentali per raggiungere lo scopo che si prefissa. Istituire la Giornata del formatore senza prevedere le necessarie risorse economiche per avviare su tutto il territorio italiano momenti di confronto e di valorizzazione rischia di far diventare questa giornata, il 14 settembre di ogni anno, un momento vuoto, forse utile per un comunicato stampa, ma di scarso valore per sostenere ed aiutare chi ogni giorno fa formazione nel nostro Paese. In altri termini, non si possono pensare le leggi tanto per fare, senza assicurare che ciò che si prevede possa poi effettivamente essere realizzato. In questo caso, lasciatemi dire ed osservare come sia proprio sbagliato ed assurdo pensare di privare delle risorse necessarie il bilancio dell'istruzione e della formazione (questo prevede la legge) per organizzare manifestazioni nella Giornata del formatore. Non ci siamo, signor Presidente, ed è per questo - lo annuncio prima di entrare nel merito dei nostri dubbi e delle nostre perplessità - che, così come abbiamo fatto in Commissione, anche oggi in Aula ci asterremo nel voto finale. Abbiamo posto anche un'altra questione, attraverso i nostri emendamenti in Commissione, che è per noi sostanziale e non solo etimologica. Avevamo infatti chiesto ai colleghi e alle colleghe di maggioranza di trasformare questa ricorrenza nella giornata dell'educatore. C'è una ragione precisa alla base delle nostre richieste, ancora una volta rigettate *in toto* dalla maggioranza, che discende dalla profonda diversità dei due concetti. Formazione ed educazione non sono la stessa cosa, è evidente. Senza dubbio, l'educazione è il concetto universale che questo Parlamento deve difendere e valorizzare. Prendendo a prestito le parole del filosofo Umberto Galimberti, voglio ricordare che abbiamo bisogno di una scuola che sappia educare, perché l'educazione porta con sé un di più rispetto all'istruzione: significa prendersi cura anche del lato emotivo, sentimentale valoriale. *Educere* significa trarre fuori, tirare fuori ciò che sta dentro; dal giovane bisogna saper estrarre qualcosa. Educare, infine, non significa solo formare, ma anche trasmettere valori fondamentali: si pensi a quelli della cittadinanza, dell'etica e della legalità che consentono di far crescere donne e uomini capaci di essere pienamente inseriti dentro la nostra società. È un punto fondamentale - lo voglio sottolineare - perché tutta la comunità educante rappresenta forse il pilastro fondamentale per il nostro Paese, il punto di partenza per costruire il futuro dell'Italia. un pilastro che questo Governo e la maggioranza parlamentare stanno mettendo in crisi. Sin dall'inizio avete ignorato i problemi che riguardano le nostre scuole, le nostre università e i luoghi della formazione. Li avete ignorati ed è stato fatto anche peggio, perché i continui tagli al mondo della scuola rischiano di produrre conseguenze drammatiche per un insegnamento di qualità, forgiato sul principio dell'eguaglianza e dei territori. Eppure basterebbe ascoltare il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che solo lunedì scorso, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, ha pronunciato parole importantissime sul valore della scuola e sulla necessità di continuare a impegnarsi per combattere l'abbandono scolastico e l'evasione scolastica, sul ruolo degli e delle insegnanti e sulla necessità di valorizzare il loro lavoro e di intervenire per migliorare i loro compensi. La scuola è movimento - ha detto ieri il Presidente - e non si ferma, è una strada su cui camminare insieme, giovani e adulti. È palestra innanzitutto di vita, per le conoscenze indispensabili che trasmette, per i valori preziosi che propone: fiducia, responsabilità, dialogo, accoglienza e rispetto. L'integrazione scolastica e la valorizzazione della comunità educante sono principi fondamentali, presenti e fondanti della nostra Costituzione. È a partire da questi concetti che dovremmo lavorare a momenti di valorizzazione delle donne e degli uomini impegnati a far crescere le nostre generazioni. Davanti al forte messaggio del presidente Mattarella, vorrei chiedere a chi oggi siede sui banchi del Governo se sente davvero di aver fatto dei passi in questa direzione. La fotografia che arriva dal mondo dell'educazione e della formazione in Italia è desolante. Il primo atto di questo Governo è stato il dimensionamento scolastico, che ha costretto le Regioni italiane a tagliare i servizi educativi sui territori, producendo un drammatico aumento delle disuguaglianze, soprattutto tra Nord e Sud. *(Applausi)*. Su questo punto però - e lo sappiamo bene in quest'Aula - avete fatto decisamente di peggio: con l'approvazione della legge sull'autonomia differenziata mettete a rischio il diritto all'istruzione sull'intero territorio nazionale. La creazione di sistemi regionali con risorse e regole differenziate penalizzerà le realtà che hanno di meno, al Nord come al Sud. Questo significa che avremo scuole di serie A e di serie B. A proposito di formatori, l'autonomia differenziata è un rischio che potrebbe ripercuotersi anche sulla qualità dell'insegnamento e sul valore dei contratti di lavoro. Aprire a nuovi contratti regionali significa solo una cosa, distruggere l'unicità della scuola pubblica italiana, che è un principio su cui si fonda anche l'unità del nostro Paese. Signor Presidente, siamo a tre mesi dalla discussione in Parlamento del disegno di legge di bilancio, ma le premesse sembrano essere decisamente preoccupanti. Anche quest'anno, come è avvenuto nel 2023, sembra chiaro che la questione della scuola e della formazione rimarrà sempre esclusa dai finanziamenti del Governo, se non addirittura penalizzata. Lo voglio dire in maniera chiara: non basta una Giornata del formatore per nascondere le gravi responsabilità che questo Governo e questa maggioranza hanno nella crisi del nostro sistema scolastico. questa battaglia di nuovo in Aula, tornando a chiedere di cancellare la precarietà degli insegnanti, chiedendo maggiori risorse per le nostre università e nuovi investimenti nei territori più complessi da governare, dove una scuola può essere anche presidio di legalità, portando avanti la battaglia contro la scellerata legge sull'autonomia differenziata. Voglio ricordare una frase di Aristotele che dovremmo scolpire sui nostri banchi, nella nostra testa e nel nostro cuore: tutti coloro che hanno meditato sull'arte di governare l'umanità si sono convinti che i destini del mondo dipendono dall'educazione della gioventù. Quante responsabilità attribuiamo al valore e al ruolo delle e degli insegnanti e quanto poco facciamo per riconoscere quel valore in termini di dignità del lavoro e del reddito?

di ogni anno sia davvero un momento strategico per pensare al futuro del nostro Paese, allora deve essere chiaro che serve un'inversione di rotta. A questa sfida non rinunciamo e la porteremo avanti in tutte le sedi, accanto alle donne e agli uomini che ogni giorno si occupano dell'educazione dei ragazzi e delle ragazze italiani. Per queste ragioni, dichiaro il voto di astensione delle senatrici e dei senatori del Gruppo Partito Democratico sul disegno di legge in discussione.

oggi dalla sede redigente un disegno di legge di grande rilevanza, sul quale mi auguro ci sarà il più ampio consenso da parte dei colleghi di tutte le forze politiche: l'istituzione della Giornata nazionale del formatore. Il 14 settembre, che per il 2024 è appena passato, sarà celebrato il sistema educativo a 360 gradi. La data scelta ovviamente non è casuale, visto che è proprio nel mese di settembre che avviene l'avvio dell'anno scolastico e della formazione professionale. Questa iniziativa rappresenta un riconoscimento fondamentale per una figura professionale che svolge un ruolo cruciale nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei nostri ragazzi e dei cittadini. ci si forma fin da piccoli e lo si può fare per tutta la vita; la formazione non ha una data di scadenza. Il formatore è colui che, con dedizione e competenza, contribuisce alla crescita personale e professionale di individui di tutte le età. In un mondo in continua evoluzione, dove le competenze richieste dal mercato del lavoro cambiano rapidamente, il ruolo del formatore diventa sempre più centrale e la sua capacità di adattarsi e innovare è essenziale per garantire che le nostre risorse umane siano sempre all'altezza delle sfide globali. Questo disegno di legge è, al contempo, un impegno che va incontro a quanto varato dal Consiglio dell'Unione europea nelle sue conclusioni sui docenti e formatori del futuro del 9 giugno 2020. Ci si ricorda come l'istruzione e la formazione, oltre a plasmare l'umanità e promuovere la trasformazione sia delle persone, che della società, rivestono importanza per la partecipazione dei cittadini a livello sociale, economico, democratico e culturale, nonché per la crescita, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la prosperità per l'intera Unione. È quindi fondamentale che un'istruzione e una formazione di qualità, pertinenti, inclusive ed eque non solo offrano ai cittadini conoscenze, capacità e competenze in linea con gli sviluppi attuali e futuri, ma ne plasmino anche gli atteggiamenti, i valori e i comportamenti, consentendo loro di progredire sul piano professionale e personale e di essere partecipanti attivi e responsabili della società. L'istituzione di una Giornata nazionale dedicata ai formatori non è solo un atto simbolico e un riconoscimento in un certo senso dovuto, ma un impegno concreto a valorizzare e sostenere questa professione. È un'opportunità per riflettere sull'importanza della formazione continua e per promuovere una cultura dell'apprendimento permanente. Tuttavia, è importante sottolineare che per rendere questa giornata veramente efficace è necessario accompagnarla con misure concrete. Per questo mi auguro che Regioni, Province e Comuni, per quanto possibile, incentivino anche le comunità stesse a mettere in campo e sostenere le iniziative formative adeguate per garantire che i formatori abbiano accesso a strumenti e metodologie all'avanguardia. Per quanto detto e per molti altri motivi che ogni giorno i cittadini vedono e riconoscono a chi svolge questa professione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Credo fermamente che questa proposta di legge rappresenti un passo avanti significativo per il settore. Invito tutti i colleghi a sostenere questa iniziativa affinché possiamo insieme riconoscere e valorizzare il lavoro prezioso dei formatori.

questa interpellanza con procedimento abbreviato sull'impatto sui conti pubblici derivanti dall'attuazione dell'autonomia differenziata è un atto di sindacato ispettivo condiviso da tutti i Gruppi parlamentari di opposizione. Lo sottolineo perché la risposta che arriva due mesi dopo, signor Ministro, poteva probabilmente arrivare almeno un mese e mezzo prima; avremmo rispettato il Regolamento del Senato le opposizioni avrebbero avuto le informazioni, che speriamo di ottenere oggi da lei, per poter costruire un confronto ancora più costruttivo sui temi rilevanti e molto delicati che le riprospettiamo. Signor ministro Giorgetti, noi abbiamo sottolineato in questa interpellanza che il disegno di legge Calderoli non attua tutto il Titolo V della Costituzione, ma un solo comma dell'articolo 116, e non rispetta quindi l'idea di fondo che abbiamo richiamato riportando i passaggi dell'articolo 119 della Costituzione in termini di coordinamento della finanza pubblica, che resta scolpita rigorosamente dentro le responsabilità dello Stato centrale. Il disegno di legge Calderoli, come è noto, è a invarianza di spesa (non c'è un centesimo, non c'è un euro), e non c'entra nulla con l'accordo unitario fatto nel 2020 in Conferenza Stato-Regioni e in Conferenza unificata. Signor Ministro, lo sottolineiamo perché gli accordi del 2020, al tempo del Governo Conte II, furono fatti preventivamente con le Regioni di qualsiasi colore politico e con gli enti locali (Città metropolitane, Comuni e Province) di ogni colore politico. L'impianto generale della legge quadro prevedeva che fosse lo Stato centrale a garantire prima i modelli di perequazione: da qui la norma

comune e condiviso da tutte le Regioni di centrosinistra e di centrodestra e da tutti gli enti locali, dovevano diventare 50 solo per la parte di perequazione infrastrutturale. Lo dico qui alle colleghe e ai colleghi delle Regioni a statuto speciale: quel fondo di perequazione infrastrutturale toccava anche le Regioni a statuto speciale, che non sono toccate dall'attuazione dell'articolo 116 comma 3 che, come sapete, riguarda le Regioni a statuto ordinario. Lo dico perché coloro - soprattutto i colleghi delle autonomie - che si sono fatti prendere dalle rassicurazioni devono sapere che non c'è più quella perequazione infrastrutturale. C'è un effetto di *spillover* fisiologico, quando si fa un accordo come quello che è stato fatto, che inevitabilmente incide anche sulle Regioni non coinvolte. Ribadiamo qui una volta per tutte che una cosa è la specialità, che riguarda solo cinque Regioni del nostro ordinamento, e un'altra è la differenziazione, che è l'oggetto di un disegno di legge capestro che avete approvato per lo scambio politico che abbiamo più volte denunciato. In base a questo, signor Ministro dell'economia, noi le chiediamo che cosa il Governo ha intenzione di rispondere al Presidente della Regione Veneto che, con lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri,

quindi un orizzonte che va oltre la vita di questa legislatura, presumibilmente e auspicabilmente anche di questo Governo (speriamo non oltre le nostre vite, perché auguro a tutti noi

hanno il limite - appunto - di non considerare l'impatto di quattro dei cespiti di uscita più importanti che incidono sul bilancio delle Regioni per quasi il 95-96 se ne spostiamo solo uno, il principio di coordinamento di finanza pubblica non viene più garantito. Mi riferisco al trasporto pubblico locale, alla sanità e ribadiamo che i LEA non c'entrano nulla con i LEP e le modalità di definizione dei LEA non c'entrano nulla con i LEP, perché hanno cristallizzato le diseguaglianze. E a chi dice che stiamo già male ed è colpa dello Stato centrale, rispondo che non è così: stiamo già male perché i LEA sono incoerenti e molte Regioni li contestano da anni; ma, siccome non c'è alcun luogo in cui ci si sieda per trovare delle soluzioni e siccome non ci sono risorse, non si fa ridistribuzione. Quindi, ci ritroviamo Regioni con lo stesso numero di abitanti che hanno tra le 600 e le 900 unità in meno tra gli operatori sanitari o un modello di prevenzione territoriale diverso e diversificato. Ma non è di questo che vogliamo parlare in questa interpellanza, signor ministro Giorgetti. Oltre a ricordare la rottura dell'unità delle Conferenze che c'era e non c'è più - perché il ministro Calderoli ha preferito partire dal Consiglio dei ministri anziché dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza unificata, salvo tornarci dopo dividendole, perché quell'unità non c'è - ci sconcerta che ieri il Governo abbia deciso di intervenire con ricorsi molto mirati sulle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna alla Corte costituzionale. Questo ricorso non fa altro che acuire uno scontro istituzionale di cui non c'era bisogno. Le Regioni hanno utilizzato un diritto che è dato loro dall'impianto costituzionale e il Governo ha deciso di acuire uno scontro che già si era consumato nelle Conferenze stesse.

nelle audizioni svolte durante il confronto sul disegno di legge Calderoli, ci ha detto testualmente (e rispetto a questo vorremmo «Il trasferimento delle nuove funzioni alle Regioni comporta la devoluzione di una quota di gettito erariale potenzialmente significativa e, contestualmente, la perdita di controllo da parte del Governo centrale di settori rilevanti della spesa pubblica. Tutte le Regioni dovrebbero contribuire alla sostenibilità dei conti e al rispetto dei vincoli di bilancio costituzionali previsti all'articolo 81 e all'articolo 97 della Costituzione, oltre che dei vincoli europei». Signor Ministro, noi vorremmo

possa proseguire la sua vita. È evidente che, senza un fondo di perequazione non solo sulle infrastrutture - come avevamo fatto nel 2020 - ma anche e soprattutto sui servizi, in particolar modo

Sottraendo allo Stato centrale anche soltanto un decimo delle entrate tributarie, le entrate complessive si ridurrebbero di circa 61 miliardi. È evidente che non tiene tiene e che non è possibile ipotizzare modelli redistributivi basati sui residui fiscali. Vista la richiesta del presidente Zaia di quelle nuove materie, signor Ministro chiarisse che non ci sono residui fiscali, ma non ci sono nemmeno le risorse per le materie non LEP. Ricordo alle colleghe e ai colleghi della maggioranza che il PIL delle Regioni del Centro-Nord è pari al 77,5 per cento di quello nazionale

di più servizi pubblici, di più trasporto pubblico locale e tutto ciò non è garantito in questo impianto. *(Applausi)*. Pertanto, signora Presidente, chiedo al Ministro dell'economia e delle finanze di chiarire una volta per tutte in quest'Aula se il disegno di legge Calderoli, che noi abbiamo definito

finanze*. Signora Presidente, nell'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interpellanti, nel rilevare che il Presidente della Regione Veneto ha formalmente chiesto l'avvio della trattativa con il Governo per ottenere le funzioni delegate alle nuove materie non LEP, che è possibile gestire in forma decentrata, nonché considerata la situazione dei conti pubblici italiani, chiedono al Ministro dell'economia delle finanze: la valutazione sui fatti esposti e se intenda attivarsi, per quanto di propria competenza, per evitare ulteriori situazioni di instabilità per le finanze pubbliche che possano derivare dall'attuazione delle proposte; se se non ritenga opportuno attivarsi per chiarire in via definitiva quale sia l'impatto atteso sui conti pubblici derivanti dall'attuazione dell'autonomia nel suo complesso e se gli effetti prodotti dalla sua attuazione siano tali da compromettere il percorso pluriennale di interventi correttivi, che sarà concordato con la Commissione europea; europea; quali siano gli effetti per la finanza pubblica dell'eventuale trasferimento delle nuove materie non LEP alla Regione Veneto e, più in generale, quale sia l'impatto per ciascuna Regione in caso di richiesta di loro trasferimento. Al riguardo, dall'esame della normativa che ha recentemente disciplinato la materia, è agevole ricavare chiare regole per la salvaguardia dei princìpi della finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio. La legge n. 86 del 2024 prevede, infatti, un articolato quadro dei limiti e delle condizioni di trasferimento delle funzioni diretto a salvaguardare l'assetto della finanza pubblica. Per il trasferimento delle funzioni concernenti i diritti civili e sociali si richiede, appunto, la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, sulla base dei costi e fabbisogni *standard* e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare i medesimi LEP sull'intero territorio nazionale. Per il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi dai LEP, lo stesso può essere effettuato secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese e comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente (articolo 4 della legge n. Pertanto, in relazione alla possibilità che si determinino situazioni di instabilità per la finanza pubblica per effetto della richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sia nelle materie LEP sia in quelle non LEP, le vigenti disposizioni rappresentano un valido presidio, poiché gli oneri connessi al trasferimento di ulteriori materie sono limitati alle risorse finanziarie, umane e strumentali già destinate al loro esercizio nel territorio della Regione che accede all'autonomia differenziata.

e la proporzionalità delle risorse destinate a ciascuna delle altre Regioni che non richiedono ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, essendo peraltro ribadito che è comunque garantita la perequazione per i territori con una minore capacità fiscale *pro capite* (articolo 9, ultimo periodo, comma 3). In altri termini, la normativa vigente salvaguarda l'assenza di ricadute negative per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dell'autonomia differenziata, nonché di ricadute a carico delle Regioni che non intendono sottoscrivere specifiche intese per l'attribuzione di ulteriori funzioni. Sulla base delle richieste contenute nella lettera della Regione Veneto, il percorso normativo prevede pertanto la ricognizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali correlate alle richieste stesse, riferibili al territorio della Regione Veneto, da considerare nell'ambito del confronto tra Governo e Regione. Conseguentemente, è da escludere la ipotizzata possibilità che le richieste regionali possano innescare ulteriori situazioni di instabilità per la finanza pubblica, stante il vincolo legislativo di trasferire le materie oggetto dell'intesa nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già destinate al loro esercizio nel territorio. Parallelamente, l'attribuzione delle materie non LEP alla Regione Veneto risulterebbe neutrale per i restanti territori regionali, nei quali l'esercizio delle stesse materie sarà garantito con le attuali risorse finanziarie, umane e strumentali, non incise in alcun modo dal trasferimento. Riguardo poi alla preoccupazione circa i potenziali effetti negativi derivanti dall'attuazione della legge n. 86 del 2024 sul percorso pluriennale di interventi correttivi che sarà concordato con la Commissione europea, si ritiene che la stessa sia infondata, considerato che diverse sono le disposizioni previste all'interno del provvedimento a tutela della finanza pubblica (appunto gli articoli 4 e 9 della citata legge n. 86) che richiamano espressamente la nuova *governance* economica europea. In particolare, l'articolo 9, comma 4, espressamente prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere, anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea. Ciò proprio al fine di non compromettere, come richiesto dagli interroganti, il percorso pluriennale di interventi correttivi, che sarà appunto concordato con la Commissione europea, ma che soprattutto sarà approvato dal Parlamento italiano. Circa infine gli specifici impatti finanziari conseguenti alla deduzione delle materie non LEP alla Regione Veneto e alle altre Regioni, appare prematura ogni valutazione, dal momento che sono in corso le istruttorie da parte delle amministrazioni competenti finalizzate a individuare con esattezza le specifiche funzioni oggetto di eventuale devoluzione. Rinvio quindi alla relazione scritta del ministro Calderoli, che invierà alle Camere prima dell'avvio dei negoziati, e alla relazione tecnica di ciascuna pre-intesa. Per concludere, onorevole Boccia, io parto da un approccio totalmente opposto al suo con riferimento al federalismo. Per lei il federalismo è fonte di maggiore spesa. Per me il federalismo è l'introduzione del principio di responsabilità a ogni livello e fonte di efficienza e di risparmio di spesa. *(Applausi)*. Condivido invece con lei Condivido invece con lei il riferimento al fatto che le Regioni, in particolare del Mezzogiorno, hanno necessità di più scuola e di più sanità. Aggiungerei però che hanno bisogno di più buona scuola e di più buona sanità. E forse l'autonomia differenziata gliele potrà garantire.

di spesa, ma deve essere il miglioramento dei servizi, magari riconducendoli a delle spese che il nostro Paese può sostenere. Conosco bene il tema della maggiore autonomia. Vengo da una Regione a Statuto speciale e ne conosco e ne conosco le opportunità, ma anche i limiti. Non credo che questa vicenda politica si possa banalmente rappresentare come uno scontro tra il Nord e il Sud, perché - l'ha detto benissimo prima il presidente Boccia vi sono aree interne di ogni Regione che hanno maggiore difficoltà a produrre ricchezza, meno servizi e meno infrastrutture. All'interno di tante Regioni del Nord vi sono intere aree che sono in sofferenza e, quindi, non è soltanto il tema del Nord contro il Sud.

a festeggiare l'autonomia come il raggiungimento di un grande obiettivo e ha fatto eventi per tutta l'estate in tutto il territorio. Ne riparleremo fra una decina d'anni quando avremo quantificato i LEP e avremo capito quanto costano le materie non LEP. Infatti, la una materia non LEP non significa che sia gratis, ma significa che devo valutare in un altro modo. Non ho un livello essenziale di prestazione, ma sicuramente ho un trasferimento di funzioni che ha un effetto sulla finanza pubblica. Quindi, caro Luca, ti faremo sapere. *(Applausi)*. Mi sembra evidente che in questo momento il Governo non è in grado di attuare la riforma per cui tanto ha festeggiato.

La necessità di agevolare e favorire l'imprenditoria, specie in tema di *start-up* e piccole e medie imprese è stata una priorità nei programmi di Governo da innumerevole tempo. Tutti i Governi e le maggioranze che si sono susseguiti hanno promesso a vario titolo misure di agevolazione e di promozione delle attività di italiane e di italiani che investono nel nostro Paese e contribuiscono alla crescita del nostro tessuto imprenditoriale. Ebbene, al di là delle tante promesse non mantenute, "dei già e dei non ancora", questa maggioranza parlamentare interviene invece con un disegno di legge che, senza se e senza ma, raccoglie il grido di difficoltà delle nostre imprese - ascoltate anche oggi all'assemblea di Confindustria ed accolte ovviamente dal nostro *premier* Meloni

che diceva - come ha fatto anche oggi il presidente di Confindustria Orsini - fare l'imprenditore in Italia è oggi un'impresa quasi eroica. Tasse altissime, una burocrazia soffocante, una giustizia ostile, infrastrutture carenti: sono tutte cose che scoraggiano gli investimenti. Oggi il nostro *premier* Meloni ha accolto questa sfida. Ecco, è proprio nel segno di tale insegnamento che si pone questo disegno di legge che ha il solo obiettivo di favorire la crescita della nostra Nazione. Entrando brevemente nel merito, cari colleghi, il provvedimento interviene in modo significativo sulla disciplina della detrazione Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentire la funzione del credito d'imposta anche in caso di detrazione più alta dell'imposta lorda a carico del contribuente. In altre parole, viene consentito al contribuente di trasformare la quota di agevolazione eccedente in credito d'imposta utilizzabile. Ancora, si esenta dall'imposizione sui redditi la somma dei proventi percepiti da persone fisiche nel caso provengano da investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio, che investono in imprese innovative. Insomma, senza entrare nel merito di tutte le singole norme che conosciamo tutti - qualcuno magari un po' comunque le abbiamo fatte proprie - non può sottacersi che si tratta di un provvedimento di immediata attuazione, che produce finalmente un taglio considerevole delle tasse per chi fa impresa e la fa in Italia, producendo ricchezza, aumentando posti di lavoro, in sostanza contribuendo al futuro dei nostri giovani *in primis* e di chiunque voglia intraprendere nel nostro Paese. Auspico che questo provvedimento trovi il pieno accordo di tutto il Parlamento e così mi è sembrato, almeno di quei parlamentari che - come noi - intendono portare avanti il mandato degli italiani sulla crescita, sullo sviluppo e sul sostegno alle imprese.

- avendo una matrice liberaldemocratica, ci poniamo da sempre al fianco delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori, cioè del sistema Italia e del sistema Paese. Signora Presidente, componenti del Governo, onorevoli colleghi, il primo provvedimento che riguarda le *start-up* innovative è del 2012, con il Governo Monti, e successivamente l'intervento forse storicamente più importante è avvenuto nella prima legge di bilancio del Governo Renzi, nel 2014, dove finalmente alle *start-up* innovative si è dato un credito d'imposta per poter sviluppare quelle imprese quelle imprese che vedono l'innovazione come elemento portante. Tutti noi sogniamo che da questi provvedimenti, in un garage italiano, avvengano quei miracoli che di solito vengono raccontati nell'imprenditoria americana, o che si scoprano grandi progetti innovativi attraverso le intuizioni di alcuni giovani. giovani. Per questo motivo, volendo rassicurare la collega Biancofiore, noi voteremo a favore, e non perché condividiamo le tesi di questo Governo, ma perché su tutto ciò che serve a fare imprenditoria noi votiamo a votiamo a favore.

stati emessi - devono avere tre anni consecutivi di bilancio positivo. Vi rendete conto che tre anni consecutivi di un bilancio positivo vogliono dire che non sei più una *start-up*, ma sei già un'azienda consolidata? Le *start-up* hanno questo di differente rispetto alle altre

nella relazione della presidente del consiglio Meloni in Confindustria, in un certo senso c'è stato un rimprovero dell'Europa troppo *green*. Ebbene, molte *start-up* sono rivolte all'ambiente, a un nuovo modo di produrre, perché i giovani forse ce l'hanno maggiormente nel DNA rispetto ad altre persone, anche soltanto della mia generazione, e quindi preistoriche.

sulle tematiche ambientali, sulle energie rinnovabili, che l'hanno come punto di riferimento. Ricordiamoci solo che il PNRR è stato portato a casa proprio perché con il 41 per cento delle risorse, in teoria con il Governo Draghi - poi questo Governo molte le ha rimandate a casa - sulla transizione ecologica c'era un intervento pesante. Noi votiamo a favore perché non vogliamo darvi l'alibi di dire che non stiamo dalla parte delle imprese. Ma questo è un provvedimento estetico,

in maniera molto meno trionfale di chi mi ha preceduto, annuncio che il nostro sarà un voto positivo, ma che, ancora una volta, questo provvedimento dimostra che non c'è una visione d'impresa del Governo per il Paese.

Essendo questo uno dei terreni in cui molti giovani investono - investono nella innovazione,

non si sono create le condizioni per dare incentivi. Si interviene, sostanzialmente, sulla questione fiscale,

di utilizzare in compensazione o in dichiarazione quel credito che altrimenti sarebbe andato perso. Quindi si dà la possibilità a tutte le *start-up* di essere parificate. Mi dispiace che non venga colto questo punto, che è fondamentale e cambia

fiscali. Cosa fa questo provvedimento sostanzialmente? Innanzitutto cerca di recuperare questo *gap*. Nell'articolo 1 si definiscono esattamente quali sono le *start-up* e quali sono i parametri per diventata una *start-up* e una PMI innovativa. Ricordo che spesso sono state create nel nostro Paese delle imprese e delle *start-up* che non avevano i requisiti, non avevano brevetti, non avevano nemmeno un dipendente e, quindi, magari venivano utilizzate in modo fittizio per ottenere delle agevolazioni. Quello che si fa è concentrare le risorse disponibili sulle reali *start-up*: questo lo fa l'articolo 1. L'articolo 2, invece, dà la possibilità tutte le *start-up* di utilizzare il credito d'imposta, anche a quelle che non hanno una capienza fiscale. Questo è un punto molto interessante che consentirà

nuove risorse che verranno impiegate grazie a questo atto logicamente avranno dei benefici maggiori rispetto alla spesa, considerando che l'innovazione rende più efficiente la pubblica amministrazione, le cure mediche, e tutti i settori ne possono beneficiare. questa chiave di sviluppo del nostro Paese logicamente vorrà dire pagare in termini di sviluppo economico, in competitività del nostro sistema e anche in termini di efficienza. Investendo Investendo in questo settore possiamo invece affrontare sicuramente meglio le sfide del futuro. Sono proprio questi gli investimenti produttivi da sostenere.

eliminando eventuali imprese fittizie e imprese che non hanno i parametri di innovazione o di *start-up*; inoltre, dà la possibilità a tutte le imprese di beneficiare degli incentivi.

di sistema fiscale. Poi l'articolo 3, in sede redigente, modifica la disciplina del patrimonio destinato amplificandone le facoltà operative, al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, delle reti e delle infrastrutture strategiche. L'articolo 4, invece, ci chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze - anche questo è un punto importante - derivanti dalle cessioni di quote di imprese innovative: nel momento in

a vantaggio delle imprese innovative, perché saranno esenti dalla tassazione delle plusvalenze. Infine, l'articolo 5 aumenta da 25 a 50 milioni il limite del patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice.

a livello nazionale. Si parla di politiche che partono dal 2012, di una crescita nel settore innovativo arrivata da diversi Governi. Siamo anche molto contenti di quello che è stato fatto nei Governi precedenti, nel Conte I e nel Conte II, dove si è spinto tantissimo in questa direzione, si è creduto molto nelle iniziative delle *start-up*

Attenzione, però: quelli non erano dati su cui adagiarsi, ma era solo un inizio, un approccio positivo, un modo di ragionare; quando ci guardiamo intorno, quando guardiamo gli altri Paesi, quelli vicini all'Italia, in particolare la Francia

intorno alla nostra. Abbiamo tracciato una strada giusta in questi anni e adesso è importante che le politiche vengano portate avanti e si lavori sulla crescita di questo settore.

è stato così. Tante delle proposte che abbiamo portato avanti all'interno della discussione sono state respinte. Abbiamo avuto un approccio estremamente costruttivo su questo provvedimento.

che chi crede nell'innovazione potesse essere premiato e anche questo non è stato recepito. Abbiamo chiesto misure più concrete per le nostre per far respirare i piccoli borghi e dare una vera e propria spinta al nostro Paese. Purtroppo non abbiamo portato a casa nulla di tutti i provvedimenti che abbiamo proposto. C'è stato un passaggio nelle due Camere, ma per l'ennesima volta siamo riusciti a incidere poco

efficiente ed efficace per raggiungere degli obiettivi, ci asteniamo perché comunque va nella giusta direzione, ma c'è davvero poca sostanza, come in tanti provvedimenti che ultimamente

che le menti brillanti del nostro Paese siano costrette a scappare continuamente e non è un provvedimento come quello in esame che fermerà l'esodo. Siamo stanchi di vedere soffocate le nostre imprese da tasse

nostro Paese questa idea possa essere realizzata e non ostacolata da burocrazia e soprattutto dai poteri forti che vediamo continuamente supportati dal corporativismo nei provvedimenti.

siamo sicuri che questi temi torneranno all'esame della nostra Commissione, dove potremo dare un forte contributo e lo faremo.

In un mondo che diventa sempre più competitivo è necessario garantire competitività al sistema Paese e quindi sostenere le nostre aziende, soprattutto quelle più innovative. dobbiamo anche renderci conto del contesto in cui siamo inseriti, in un'Europa che - ahinoi - sta perdendo competitività, anche e soprattutto per scelte banalmente ideologiche e non legate a logiche di mercato. Pensiamo a quello che sta succedendo al mercato dell'auto e alla produzione *automotive*; qui noi abbiamo veramente l'immagine di cosa non bisogna fare. Diciamo di voler puntare sull'innovazione e dall'altra parte abbiamo tutto un sistema che mette delle regole che, in via ideologica, limitano l'innovazione e puntano alla recessione. Guardiamo cosa succede ai nostri principali *competitor*. La Germania, ex locomotiva d'Europa, è sostanzialmente ferma. Ha perso i due vantaggi competitivi di fondo: l'energia a basso prezzo l'effetto delle politiche di contenimento dei salari fatte dai Governi di sinistra nei lustri precedenti hanno esaurito il proprio corso.

Noi invece abbiamo le nostre multinazionali tascabili, le nostre piccole e medie imprese, che, come motoscafi, possono cambiare rotta molto velocemente: è lì che dobbiamo puntare. L'altro nostro competitore importante, la Francia, è ormai da decenni con la bilancia commerciale in passivo. Ci insegnavano una volta, quando si studiava economia nelle scuole superiori e all'università, che la bilancia commerciale in passivo prima o poi la paghi. E la si sta pagando non solo con una ancora non chiara *governance* politica, ma soprattutto dal punto di vista economico. Quindi l'Italia, in questi frangenti, si trova in una posizione migliore. Ottima? Certo che no, perché abbiamo - ahinoi - un debito che è il doppio di quello della Germania e, quindi, paghiamo il doppio degli interessi. chiaro che, se avessimo un debito più basso, avremmo il doppio dei margini; però dal punto di vista dei fondamentali economici possiamo ancora dire la nostra, e dobbiamo dire la nostra. E possiamo farlo se, con coerenza, portiamo avanti

La pubblica amministrazione crea servizi per consentire alle imprese di creare PIL e fare buona economia. In conclusione, con questa legge noi ci muoviamo in coerenza con quelle che sono state le nostre azioni politiche. Pensiamo a quello che ha fatto la Lega negli ultimi anni, per esempio alla *flat tax* e alle detassazioni per le partite IVA e per le piccole imprese artigiane e commerciali.

un'inversione rispetto a quelle politiche di sussidi che hanno generato non solo uno sperpero enorme di risorse pubbliche, ma anche una sperequazione, perché hanno favorito soprattutto i redditi alti, con i soldi tasse pagate dai ceti medio-bassi, quindi anche dal punto di vista dell'equità. Inoltre i sussidi di carattere sociale hanno spinto a non cercare occupazione. La stretta su queste due politiche di sussidi ha portato a quello che abbiamo oggi, che è il *record* di occupazione. Siamo contenti? No: si può fare ancora di più. Però la linea è tracciata: fare l'opposto e quindi, puntare non su politiche di sussidi, ma su chi crea PIL, lavoro e sviluppo, che sono le aziende. E con questo disegno di legge noi andiamo esattamente in questa direzione. *(Applausi)*. Signor Presidente, i colleghi hanno già richiamato il fatto che la prima disciplina organica sulle *start-up*, in particolare su quelle innovative di cui il Paese si è dotato, risale al 2012, e quindi è passato più di un decennio. Quella disciplina, in realtà, ha avuto un discreto successo nel promuovere gli obiettivi che si era data, anche attraverso l'istituzione di un apposito registro dedicato alle *start-up* innovative che, nel corso del decennio, si è notevolmente popolato, passando da circa 1.400 *start-up* innovative nel 2013 a oltre 14.000 nel 2022. È chiaro che, a distanza di tanti anni, la disciplina necessitasse di una revisione. Ci saremmo aspettati un intervento di natura organica, una sorta di Start-up Act Act 2, visto che la prima norma fu battezzata Start-up Act. In realtà, la maggioranza e il Governo hanno scelto una via per intervenire e rivedere la disciplina del tutto frammentaria e disorganica.

un intervento che chiama in causa misure da affidare, nella propria implementazione, a Cassa depositi e prestiti tramite l'utilizzo del patrimonio destinato. Rispetto a queste noi non abbiamo una posizione pregiudizialmente contraria; anzi, riteniamo sia utile mobilitare tutti gli strumenti disponibili per sostenere l'ecosistema innovativo delle *start-up.* Avremmo però voluto contribuire all'arricchimento e alla discussione della misura, anche vedendoci un po' più chiaro sul pregresso. Avevamo chiesto, anche in Commissione, di utilizzare questa occasione di revisione della normativa sulle *start-up* per guardare dentro al patrimonio destinato: come era stato utilizzato e quante e quali risorse fossero ancora a disposizione di quel fondo. Tuttavia, maggioranza e Governo non hanno voluto aprire la scatola nera e non è stato possibile utilizzare questa occasione per fare degli approfondimenti e delle valutazioni di politica economica sui temi del sostegno alle imprese innovative. Ciononostante, il nostro giudizio sul provvedimento nel suo complesso non è negativo, nel senso che anche il Gruppo Partito Democratico esprimerà un voto di astensione, perché tutto quello che migliora e incentiva l'ecosistema dell'innovazione ci vede favorevolmente schierati. Riteniamo che non sia sufficiente e anche che sia contraddittorio il fatto che, mentre noi oggi approviamo una revisione

del tutto disorganiche rispetto alla necessità di unificare in un unico testo la disciplina sulle *start-up* innovative. Vorremmo che nel prossimo futuro Governo e maggioranza prestassero attenzione alla costruzione di provvedimenti non così strabici, che procedono a spizzichi e bocconi, intervenendo sulla stessa materia, ma raggruppando invece in una disciplina organica, facilmente intellegibile per operatori e investitori, tutto quello che riguarda lo stesso tema. Vi è anche un ulteriore punto su cui non è stato dato seguito all'impegno del primo Start-up Act, cioè il tema delle imprese innovative a vocazione sociale, le *start-up* ad impatto sociale, rispetto al quale noi pensiamo sia necessario un ulteriore intervento di sostegno, che non trova attenzione né in questo disegno di legge né nel disegno di legge sulla concorrenza che affronteremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Il nostro è un voto di astensione tale da segnare la disponibilità del nostro Gruppo e del nostro partito politico nei confronti di tutte le materie che riguardano le *start-up* e le *start-up* innovative. Speriamo che ci sia l'occasione per riprendere insieme alla maggioranza e al Governo il filo di un ragionamento un po' più organico di questi interventi, interventi, spesso frammentari e alcune volte addirittura strabici, che in questi mesi abbiamo dovuto esaminare e approvare su temi analoghi, soprattutto su temi di natura economica e di politica economica.

se c'è una caratteristica che più di ogni altra nel corso della storia ha rappresentato l'emblema di italianità e ancora oggi rende illustre il nostro Paese agli occhi del mondo, essa è senza dubbio la creatività, ovvero quell'arte del partire da quanto si ha a disposizione per rivoluzionarlo ed esternare un capolavoro. Spesso si parte da molto poco, si ha a disposizione pochissimo. La creatività non è una fredda e meccanica presa di un materiale per renderlo funzionale, ma significa saper coniugare questa efficienza, certamente necessaria, almeno per noi, con la bellezza che, in termini meramente pratici, può sembrare superflua, ma che, al contrario, costituisce un essenziale valore aggiunto, il vero sale di ogni cosa. L'Italia in questo è stata e tutt'oggi è maestra, non solo nelle tradizionali forme dell'arte espressiva, ma nella vera e propria arte di vita applicata ad ogni campo della quotidianità. Questa forma di ingegno si traduce nell'importante capacità imprenditoriale che si può dire essere quasi innata nel popolo italiano; arte anch'essa alla pari di tutte le altre, arte che va incentivata, tutelata e messa nelle condizioni di poter dare vita a piccoli capolavori. Questo è esattamente l'obiettivo della misura che ci apprestiamo a votare, ovvero il supporto alla creazione e alla crescita di *start-up* e PMI dal carattere innovativo, opere generalmente frutto di molto studio, notevole impegno e grande creatività. In primo luogo la norma definisce l'ambito di applicazione delle misure agevolative previste, facendo riferimento a due leggi precedenti. Le ripeto perché mi sembra che non siano state

l'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative. A tal proposito mi preme solo rammentare che entrambe le norme prevedono che, al fine di ricadere nelle due definizioni configurate, la società deve possedere dei requisiti seri, ad ad esempio, un determinato volume di spese in ricerca, sviluppo e innovazione, un minimo del 15 per cento, o una determinata percentuale della forza di lavoro complessiva dell'impiego, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, di dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori in Italia o all'estero oppure di personale in possesso di laurea magistrale o, infine, la titolarità di un brevetto, cioè una cosa da loro inventata. In altri termini, incentivando e tutelando questo tipo di società, si tutela il futuro della nostra Italia, si incentivano i giovani, le nostre eccellenze, offrendo loro un'altra possibile strada rispetto al trasferimento all'estero. Si promuove lo sviluppo tecnologico essenziale per far rimanere l'Italia al passo con le altre potenze globali. Attraverso due articoli si interviene, da un lato, sulla disciplina delle detrazioni Irpef, ampliandone lo scopo e prevedendo che, anche in caso di incapienza del contribuente, ne sia consentita la fruizione per gli investimenti tramite trasformazione di un credito d'imposta; dall'altro, si esentano dall'imposizione, a determinate condizioni, le plusvalenze che vengono conseguite o da chi cede le partecipazioni al capitale di questo tipo di imprese, o da chi le plusvalenze ottenute le reinveste nelle stesse. Ciò sembrerà poco, o addirittura irrilevante agli occhi dei contestatori seriali (e ne leggiamo tanti), ma in questo modo si consente un mercato più rapido delle partecipazioni e la possibilità che queste aumentino di valore molto rapidamente. Si agevola altresì anche il normale piccolo contribuente, che magari decide di investire, ad esempio, nel sogno di un gruppetto di giovani locali, o del vicino di casa. Si ha così anche l'effetto indiretto di rafforzamento dei legami intracomunitari, nonché di quelli intergenerazionali. Incentivare questo tipo di imprese significa dunque sostenere la creatività, di cui siamo estremamente ricchi e che costituisce una delle materie prime più importanti che abbiamo come Stato nazionale. Significa aiutare i giovani meritevoli e sostenerli nella realizzazione dei propri progetti: non solo sogni, ma progetti concreti. Significa scegliere verso quale tipo di futuro si intende proseguire. È per questo che la misura al voto non è che una parte di un disegno politico più ampio, che va dalla riforma fiscale ai provvedimenti in materia di concorrenza, o in materia famiglia: un disegno coerente e con il chiaro obiettivo di valorizzare realmente il diritto all'iniziativa imprenditoriale, il quale non è altro che una sfumatura del diritto fondamentale alla realizzazione personale. Il genio imprenditoriale italiano è ciò che nel tempo ci ha reso quello che siamo ed è nostro dovere continuare a stimolarlo. Oggi leggiamo nei dati pubblicati dall'Organizzazione mondiale del commercio che l'Italia, la nostra Italia, supera il Giappone e raggiunge lo storico risultato di quinta potenza mondiale nelle esportazioni, seconda a Stati come la Cina o gli Stati Uniti, dimostrando la grande forza attrattiva della nostra Nazione, del nostro *made in Italy* e le ottime politiche in materia internazionale, anche europea, portate portate avanti in questi due anni dal Governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni. Signora Presidente, come abbiamo dimostrato più volte, a noi gli sprechi non piacciono. Noi siamo consapevoli che ogni misura che richiede fondi deve essere un investimento e come tale produttiva, perché tali fondi provengono direttamente dalle tasche dei contribuenti italiani e, per il rispetto che ad essi dobbiamo, con forza rigettiamo ogni allocazione di denaro non pensata, o meglio pensata male, che invece a qualcuno è piaciuto fare in passato. Presidente, noi alle rotelle dei banchi, di cui spero si occupi qualche neocommissario, preferiamo le rotelle dei meccanismi cerebrali delle teste dei nostri cittadini, dei nostri giovani sempre attivi e funzionanti nei secoli.

onorevoli colleghi, si giunge oggi all'esame di quest'Assemblea del disegno di legge n. 1151, approvato in prima lettura dalla 7ª Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, di cui la 7ª Commissione permanente ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 30 luglio, senza introdurre alcuna modifica. si compone di due articoli. L'articolo 1 è composto da due commi e stanzia un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Com'è noto, il Macerata Opera Festival è una delle più importanti rassegne liriche italiane, pertanto uno dei principali eventi per la valorizzazione e la diffusione della cultura musicale, che risulta così meritevole di un sostegno pubblico straordinario. L'articolo 1, sempre al comma 1, novella la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei *festival* musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale. Nello specifico, incide sull'articolo 2 di tale legge, inserendo l'associazione tra i destinatari dei contributi straordinari ivi previsti. Invece, il comma 2 subordina la concessione del contributo alla previsione, nello statuto dell'associazione beneficiaria, della nomina di un componente del consiglio di amministrazione da parte del Ministero della cultura. L'articolo 2, invece, prevede che agli oneri suddetti, pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

non perché siamo contrari *a priori* a questo provvedimento, anche perché riguarda un bene importante, culturalmente riconosciuto a livello nazionale. Tutte le

bisogna anticipare il fatto che il Macerata Opera Festival è un punto di riferimento nella cultura del nostro Paese, un luogo meraviglioso, dove da anni viene fatta opera lirica in un contesto assolutamente straordinario. per quanto ci riguarda, ogni volta che si trovano dei finanziamenti da portare all'interno del comparto culturale, questa ci pare una buona notizia. Vi sono, però, alcuni passaggi in questo provvedimento che non ci convincono. Non ci convince, ad esempio, il comma 2 dell'articolo 1. Si stanzia un importo senza che si sia spiegato alla Commissione cultura del Senato perché quell'importo e senza un progetto. C'è un C'è un importo, ma non c'è una spiegazione di quell'importo. Al comma 2 dell'articolo 1 si subordina quel finanziamento al fatto che il Ministero della cultura possa inserire un consigliere d'amministrazione all'interno della Fondazione. Questo oggettivamente è un po' strano e crea anche un precedente piuttosto pericoloso, perché non ci pare che il Governo possa mettere delle condizioni da questo punto di vista: o serve il finanziamento e quindi lo si dà, oppure non serve e non lo si dà; non è che lo si dà a condizione che il Ministero della cultura metta una figura all'interno del consiglio di amministrazione. non avendo alcun tipo di informazione su questo finanziamento e su come verrà utilizzato, abbiamo detto: se volete inserire una figura nel consiglio di amministrazione, allora specifichiamo che non venga retribuita. Nelle fondazioni liriche, ad esempio, non vengono retribuiti i consiglieri, quindi facciamo che questa figura che il Ministero vuole inserire come condizione per poter ricevere quel finanziamento non sia retribuita. Ve lo abbiamo chiesto con un emendamento e lo avete bocciato; bocciandolo state dicendo che questa figura che volete inserire all'interno del consiglio d'amministrazione sarà pagata. Faccio una domanda: se questa persona avrà uno stipendio di 400.000 euro, vuol dire che oggi stiamo finanziando una nuova poltrona dentro la Fondazione senza sapere quei soldi che fine faranno? Che gestione dei soldi pubblici è questa?

una serie di questioni poco chiare che invece vanno chiarite. Nella nostra Commissione arrivano troppo spesso richieste di finanziamento di cui non si capisce il motivo e il criterio. Devo dire che con i miei colleghi in Commissione - ringrazio in particolare il senatore Castiello - abbiamo tentato di portare avanti un principio, che è quello di decidere i requisiti attraverso i quali si può avere accesso a un finanziamento pubblico; dopodiché, in base a tali requisiti, si si va nella direzione di dare i finanziamenti a chi li possiede. In assenza di requisiti, non vorremmo che la condizione per avere dei finanziamenti da questo Governo sia avere degli amici nel Governo avere il santo in paradiso, il senatore del tuo territorio che porta un documento in Commissione e ti fa avere il finanziamento: questa è roba da Prima Repubblica. Quello che è successo ultimamente nel Ministero della cultura vi dovrebbe un minimo far cambiare rotta *(Applausi)* e non continuare ad andare avanti nella stessa direzione, che non ha portato esattamente lustro né al nostro Paese né a questo Governo (e non è la prima volta che accade). Abbiamo un finanziamento ad una Fondazione meritevole (e questo ci sta), ma le modalità con cui si vuol dare questo finanziamento sono torbide, non sono chiare e trasparenti:

Non c'è alcuna specifica per cui questo Governo dia finanziamenti alle fondazioni culturali e questo è grave perché alimenta un sistema che non è trasparente. Questo non è l'unico problema che c'è al momento, volendo fare un ragionamento più ampio rispetto al Ministero della cultura. È chiaro che si vive un momento particolare, soprattutto per questo Ministero: è cambiato il Ministro

Stiamo facendo proposte da due anni: abbiamo fatto una proposta per ripristinare i corpi di ballo stabili all'interno delle fondazioni; il 21 marzo 2024 ho interrogato il ministro Sangiuliano, il quale mi rispose in modo vago; il giorno successivo, il 22 marzo, uscita una nota del sottosegretario Mazzi che diceva: vogliamo aprire dei nuovi corpi di ballo, ripercorrendo esattamente il nostro disegno di legge. A noi va bene se ci copiate *(Applausi)*, ma rispettate l'*iter* parlamentare; non è possibile ignorare i parlamentari e poi fare i comunicati stampa. Su questo quindi non si sa cosa si voglia fare. Abbiamo una proposta sugli asili musicali. Gli asili musicali sono di destra o di sinistra? È una bella proposta quella di avvicinare i bambini fin da subito all'arte, alla bellezza, alla cultura; facciamolo, lavoriamoci insieme, con criteri trasparenti e aperti. Della natura giuridica delle fondazioni liriche parliamo da due anni, il Ministro aveva detto che anche lui era per parlare

ma con quale criterio? Questa cosa va specificata, perché questi sono soldi pubblici e non si possono utilizzare attraverso telefonate tra Sottosegretari e alcune fondazioni che promettono finanziamenti extra-FUS. Ad oggi, l'unica riforma che ha fatto il Governo sulla cultura è quella di cambiare il nome del FUS, che non è esattamente un grande risultato, da Fondo unico per lo spettacolo a Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ma non bisognava cambiare il nome, bisognava metterci nuove economie, fare nuovi investimenti, perché cambiare il nome non è una svolta.

una mano ad una fondazione assolutamente meritevole, ma i criteri e le modalità con cui lo avete portato avanti non possono far sì che si voti a favore di un importo di cui non si sa niente, 400.000 euro di cui non si conosce la motivazione,

il Macerata Opera Festival si è conquistato nel corso degli anni un posto di assoluto rilievo nella cultura non solo italiana. L'evento, che si svolge ogni anno nei mesi estivi, richiama nella città marchigiana turisti e melomani da ogni parte del mondo. Oggi si può dire che esso sia uno degli appuntamenti più importanti e attesi dal mondo della lirica. Grandissimi artisti, infatti, hanno solcato il palcoscenico del Festival, da Luciano Pavarotti a Placido Domingo, da José Carreras a Katia Ricciarelli. A fare da cornice alle opere rappresentate è lo Sferisterio, il monumentale e imponente teatro all'aperto a ridosso del centro storico di Macerata, uno dei maggiori esempi dell'architettura neoclassica italiana. Realizzato due secoli fa, aperto al pubblico nel 1829, lo Sferisterio contribuisce non poco a dare ulteriore prestigio e spessore al Festival. Già solo da questi pochi cenni, credo che sia quanto mai opportuno, anzi direi necessario e doveroso che la politica sostenga con forza il Macerata Opera Festival. I motivi sono molteplici: prima di tutto, occorre non disperdere, anzi consolidare l'eccellente lavoro fin qui svolto, permettendo agli organizzatori di garantire, anche per le prossime edizioni, il livello qualitativo raggiunto dalla manifestazione e, più in generale, il nostro sostegno è poi fondamentale per dare corpo e sostanza all'obiettivo che ci siamo proposti di promuovere e valorizzare il nostro patrimonio culturale e civile, l'espressione in ogni sua forma del bello che identifica il nostro Paese nel mondo. L'opera, come si sa, è un'eccellenza tipicamente italiana, si può dire che essa sia il contributo più importante o comunque più riconosciuto che il nostro Paese ha dato alla cultura moderna. Il termine stesso «opera» è stato assunto senza essere tradotto in tutte le principali lingue e non è altresì un caso che l'Italia possegga il maggior numero di teatri lirici al mondo. L'Italia, insomma, ha donato al mondo stesso le opere ancora oggi più rappresentate, grazie al genio e alla maestria dei propri compositori. Si può perciò dire che nessuna forma artistica rappresenti meglio il genio italico, cioè la tradizione e l'identità stessa del nostro Paese. Sarebbe però errato considerare l'opera solo un bene immateriale, perché essa unisce non solo teatro e canto, ma anche lavoro culturale e lavoro tecnico; la messa in scena impegna professionisti ed esperti dei più diversi settori. L'opera esalta quindi, come forse nessun'altra forma artistica, quel saper fare che è proprio della più alta artigianalità italiana; il lavoro di squadra, l'armonia e la ricerca della perfezione richiamano direttamente la tradizione delle scuole artistiche e delle botteghe rinascimentali. Per tutte queste ragioni, l'anno scorso l'UNESCO ha proclamato il canto lirico italiano come patrimonio dell'umanità, un riconoscimento di assoluto valore che ci impegna ancora più nella sua difesa. Bene, quindi, ha fatto l'onorevole Latini della Lega e i colleghi firmatari del disegno di legge della Camera ad accogliere le proposte di sostegno che venivano dal territorio, *in primis* dal sindaco di Macerata Sandro Parcaroli.

per motivare il voto di astensione del Gruppo Partito Democratico. Già altri colleghi hanno ricordato l'importanza del Macerata opera festival, un'eccellenza riconosciuta, organizzata dall'Associazione Arena Sferisterio. d'eccellenza, ma anche di un luogo particolarissimo, che rappresenta davvero uno dei più importanti esempi di architettura neoclassica. Vorrei anche dire che quello che noi oggi stiamo votando è un testo unificato, frutto anche di una proposta di legge del Partito Democratico, a prima firma dell'onorevole Manzi.

una modifica statutaria che preveda nel consiglio di amministrazione dell'associazione (perché stiamo parlando di un'associazione) un componente nominato dal Ministro della cultura sia un pericoloso precedente,

Ciò ne lede profondamente l'autonomia e pertanto, solo per questo motivo, ma profondamente consapevoli del valore dell'iniziativa che andiamo a sostenere, dichiaro il voto di astensione del Partito Democratico.

Fu inaugurato nel 1829, finanziato dai cosiddetti 100 consorti, cittadini maceratesi benestanti che volevano una struttura per il gioco della palla col bracciale, uno sport in voga nella metà dell'Ottocento. Questo particolare gioco richiedeva un ampio spazio aperto, delimitato da pareti contro le quali la palla poteva rimbalzare. Lo Sferisterio di Macerata fu progettato appositamente per soddisfare queste esigenze, con un imponente muro di diciotto metri di altezza e ottantotto di lunghezza, costruito aderente alle antiche mura della città. Oltre al gioco della palla col bracciale, che è tuttora presente in altre località delle Marche, lo Sferisterio ospitò anche spettacoli pubblici, come celebrazioni di feste, l'organizzazione di giostre, parate equestri, manifestazioni politiche e sportive. L'armonia interna degli spazi, il colonnato neoclassico, l'alto muro rettilineo e la grande arena aperta centrale suggeriscono, nel 1921, una sfida ambiziosa. Il conte Pier Alberto Conti sogna di organizzare un'opera lirica a Macerata, «Aida» di Giuseppe Verdi. Lo Sferisterio viene rinnovato con la costruzione di un ampio palcoscenico e l'apertura di una porta centrale, che è tuttora utilizzata, sul maestoso muro. Il 27 luglio 1921, di fronte a 10.000 persone giunte da tutta Italia, va in scena la prima rappresentazione: è un grande successo, visto da circa 70.000 persone nelle 17 serate di repliche. Questo evento segnò l'inizio di una nuova era per lo Sferisterio, trasformandolo in un importante polo per la musica e l'opera. La sospensione delle attività imposta dalla guerra fu interrotta solo per il memorabile concerto tenuto nel 1927, quando si esibì nell'anfiteatro il recanatese Beniamino Gigli, in un concerto vocale e strumentale accompagnato dal maestro Amilcare Zanella, uno fra i più grandi direttori d'orchestra dell'epoca. Il successo fu tale che il ricordo ancora si perpetua nell'iscrizione celebrativa posta all'ingresso principale. Soltanto nel 1967 riprende l'attività lirica dello Sferisterio, dopo l'interruzione dovuta alla Seconda guerra mondiale. Dal 1967 richiama pubblico da tutto il mondo per l'unicità delle sue proposte artistiche e per il fascino del luogo. Prestigiosi gli artisti che si sono esibiti sul palco, a partire da Mario Del Monaco, che ha interpretato Otello, l'opera che ha riaperto lo Sferisterio. Voglio citare solo alcuni di coloro che hanno calcato quel palco, da Katia Ricciarelli a Placido Domingo, da José Carreras a Franco Corelli, da Rudolf Nureyev a Luciano Pavarotti, che lo definì il più affascinante teatro all'aperto che avesse mai visto. Oggi, con l'acustica naturale, più di 3.000 posti, 104 palchi e un palcoscenico di dimensioni notevoli, l'Arena Sferisterio è considerato uno dei principali teatri all'aperto d'Italia, secondo solo all'Arena di Verona per rilevanza e fama. Nelle stagioni estive ospita infatti il Festival dell'opera di Macerata, con il grande contributo dei professionisti della FORM, l'orchestra filarmonica marchigiana, oltre ad eventi musicali complementari al cartellone lirico. Voglio ricordare il Musicultura Festival, oltre a vari concerti di musica leggera e jazz. Viene definita a ragione un'officina delle meraviglie. Voglio ricordare anche la valenza sociale dello Sferisterio, con il progetto InclusivOpera che da sedici anni fa sì che tutte le opere siano accessibili al pubblico cieco o ipovedente, con audiodescrizioni e audiointroduzioni, sia in italiano che in inglese. In abbinamento a ciascuna opera vengono inoltre offerti percorsi partecipativi, inclusivi e multisensoriali, anche in lingua italiana dei segni (LIS), guidati da giovani con disabilità sensoriale. Al pubblico sordo e ipoudente viene inoltre offerto un servizio di ascolto assistito, oltre ai sopratitoli in italiano e in inglese per tutte le recite del Festival. Grazie a questo di disegno di legge voglio rispondere a chi non si è convinto a dare un voto favorevole, sperando che possa cambiare idea in questi ultimi minuti, voglio specificare che a decorrere da quest'anno, che ha coinciso con il sessantesimo del Macerata Opera Festival, sarà previsto un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione, per l'organizzazione appunto del MOF, attraverso una modifica alla legge 2 dicembre 2012, n. 238, che prevede appunto il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani, prevedendo altresì la nomina di un componente del consiglio di amministrazione da parte del Ministero della cultura. Voglio anche ricordare come, proprio lo scorso anno, l'UNESCO abbia

di Macerata, per l'Italia, ma anche nel mondo della lirica. Presidente, colleghi, da marchigiana ed esponente della Provincia di Macerata vi ho raccontato, con l'orgoglio di appartenere a questa terra, una delle meraviglie che ma anche che si offre, aprendosi al mondo ogni anno attraverso l'opera, la musica e le arti. Ciò che ci apprestiamo ad approvare oggi è un riconoscimento che sottolinea ulteriormente il valore dello Sferisterio nel panorama italiano e internazionale e l'importanza che ricopre per noi il sostegno alla cultura. Se parliamo di cultura, ma manchiamo di sostenerla nel momento del bisogno, non siamo coerenti con ciò che portiamo avanti nel nostro impegno e attraverso le nostre parole.

Signora Presidente, questa mattina si è spento a Palermo Totò Schillaci, che ha perso la sua sfida contro il cancro. Di sfide lui ne ha però vinte tantissime, calcando i campi di calcio più importanti. come capocannoniere. È stato lui a portare la magia in quelle notti del 1990, in cui ha vinto il titolo di capocannoniere dei Mondiali e di miglior giocatore. Ha sfiorato anche il Pallone d'oro, arrivando secondo. C'è una curiosità: dopo le notti magiche di Italia '90 le parole italiane più conosciute e pronunciate nel resto del mondo erano pizza e Schillaci.

perché è stato un esempio di riscatto per tutta la città di Palermo. È stato l'orgoglio della città di Palermo ed è stato un esempio per i giovani perché forse non tutti sanno che, all'inizio della sua carriera, a Messina, ha subito ben due interventi al menisco,

che oggi piange il suo campione. Sono veramente emozionata perché ero piccola quando gli vedevo sgranare gli occhi in quelle notti magiche e il suo esempio e il suo ricordo rimarranno sempre con noi.

passato gran parte della sua vita a giocare in serie B. Inoltre, come è stato detto, è stato un siciliano che ha giocato molto in Sicilia ed è stato molto attivo nelle attività che riguardano la città di Palermo.

Totò Schillaci è stato molto attivo nelle attività sociali, nell'aiutare una squadra di calcio di rifugiati e nel fare del riscatto e della solidarietà il momento esemplare il momento esemplare della sua vita non solo da campione, ma anche da cittadino. Noi oggi lo ricordiamo come un grande campione, ma anche come un grande esempio per i campioni di domani e per i cittadini tutti.

che dalla periferia ha dimostrato che si può sfidare il mondo. Signora Presidente, Totò Schillaci è uno degli eroi dei mondiali di Italia '90 che hanno fatto grande il nostro calcio e il nostro Paese. Oltre a essere titolare del Palermo, come molti hanno ricordato, da juventina mi piace ricordarlo nella mia Juventus, quella di Roberto Baggio e di Totò Schillaci, dove i gemelli del gol tornavano ad essere insieme. Con la Juventus ha vinto una Coppa Italia e una Coppa UEFA,

uno di quei protagonisti del calcio operaio che diventavano improvvisamente importanti, tanto da essere uno dei primi a varcare i Paesi stranieri. Ricordo infatti che finì la sua carriera

Signora Presidente, la notizia era ancora calda questa mattina e già si leggevano, scorrendo le pagine dei *social*, tanti messaggi di di affetto nei confronti di un grande sportivo che ha segnato la storia del nostro calcio italiano, ma anche del mondo. Tra i tanti commenti che ho letto questa mattina, uno di quelli che più mi hanno colpito e mi sono

Presidente, onorevoli colleghi, intervengo oggi in Aula perché nelle scorse ore la mia provincia, quella di Foggia, è stata investita da una fortissima ondata di maltempo e purtroppo il capo reparto dei Vigili del fuoco, Antonio Ciccorelli, mentre era in servizio, ha perso la vita. L'auto su cui viaggiava insieme alla sua squadra è stata travolta da una piena del torrente. Il collega, Filippo Civetta, che era con lui e al quale auguriamo una pronta guarigione, è rimasto ferito. Il corpo del vigile è stato recuperato nelle prime ore del mattino dai colleghi sommozzatori. Antonio Ciccorelli aveva poco più di sessant'anni ed era prossimo alla pensione, dopo una vita di lavoro al servizio del Paese. Ai suoi familiari, ai colleghi e agli amici vanno le nostre più sentite condoglianze. un dovere ricordare il sacrificio di un uomo che ha dato la sua vita per il bene degli altri. Il suo impegno, l'altruismo e lo spirito di servizio resteranno da esempio, la sua memoria sia di conforto e ispirazione per tutti i colleghi, i familiari e gli amici. Antonio Ciccorelli è vittima del dovere. A quanti perdono la vita in servizio deve arrivare forte la nostra riconoscenza. Ogni vita persa in servizio è una perdita incolmabile per le famiglie, per le comunità e per l'intero Paese. ci sono a volte dei momenti e degli argomenti nei quali noi siamo all'opposizione e si interviene come parlamentari di opposizione. questo argomento, però, che abbiamo sollevato anche stamattina con una dichiarazione pubblica e oggi vogliamo ripetere in Aula, interveniamo come parlamentari che hanno a cuore l'interesse generale del Paese e, nel caso, la sua sicurezza. Stamattina siamo intervenuti come parlamentari del PD, membri della Commissione antimafia; qui al Senato, oltre a me, c'erano la senatrice Rando, la senatrice Valente e il senatore Mirabelli.

Poi, riportando cose che avrebbe pronunciato durante la deposizione alla procura di Perugia sul caso cosiddetto Striano-Laudati e sulle attività di dossieraggio, lo stesso Ministro della difesa si riferisce all'AISE (Agenzia contestato in più di un'occasione mancate informazioni alla Difesa, che avrebbero potuto anche creare problemi alla sicurezza nazionale. Così il Ministro della difesa dell'attuale Governo si riferisce agli apparati di sicurezza del Paese, a cui aveva contestato mancate informazioni che avrebbero potuto causare problemi alla sicurezza nazionale. È chiaro che anche l'interlocutore non è solo l'ex o l'attuale vertice dei Servizi, ma anche chi ne ha la delega: oggi ce l'ha il sottosegretario Mantovano. È uno scontro nel Governo, che però non voglio

gravi rischi per la sicurezza cibernetica del Paese (è stato anche usato il termine «colabrodo» per definirli), rischi non solo di accessi abusivi, ma di penetrazione e di hackeraggi nel sistema di sicurezza informatica del Paese e nelle banche dati, in un momento difficilissimo per la geopolitica, queste affermazioni del Ministro della difesa in carica nei confronti del suo interlocutore, che ha la delega ai servizi segreti, l'onorevole Mantovano, richiedono un immediato chiarimento, non solo, giustamente, a livello di Copasir, per le parti che devono essere secretate, né nella Commissione antimafia, dove continueremo a lavorare per fare piena luce su quel sistema di accessi abusivi; questo perché gli esecutori li conosciamo, anche gli eventuali mandanti, nell'interesse di tutti, perché lo dobbiamo fare. Abbiamo bisogno però che su questo scontro, che riguarda la sicurezza del Paese, secondo il Ministro della difesa, la presidente del Consiglio Meloni venga subito in Parlamento a riferire. *(Applausi)*. Vogliamo capire se la sicurezza del Paese è davvero stata ed è a rischio, a che punto stanno tutte le misure per evitare che alcune cose avvenute non accadano più e per essere sicuri che, in un momento come questo, il sistema Italia sia nell'assoluta sicurezza. Per questo ribadiamo, anche in Aula, la necessità che al più presto la Presidente del Consiglio venga a spiegare in Parlamento che cos'è successo tra il suo Ministro della difesa e il suo Sottosegretario con delega ai Servizi. Senatore Verini, come ben sa, questo è un argomento che può essere trattato nella Conferenza dei Capigruppo, quindi può assolutamente avanzare questa richiesta anche al suo Capogruppo.